L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato,

Onorevole Presidente, informo la S.V. che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, ha accettato le dimissioni dalla carica di Vice Ministro e di Sottosegretario di Stato per il Ministero dell'interno rassegnate dal sen. dott. Filippo BUBBICO. *F.to* Paolo GENTILONI».

il collegato fiscale rappresenta, insieme alla legge di bilancio che ci apprestiamo a esaminare nelle prossime ore, il passaggio di avvio della manovra di bilancio per l'anno in corso. Il provvedimento ci consente, allo stesso tempo, non soltanto di discutere sulle importanti misure in esso contenute, ma anche di fare un bilancio complessivo del lavoro svolto in questi anni. Il nostro Paese si trova oggi in una situazione di finanza pubblica sotto controllo e con una crescita economica che si attesta su buoni livelli. In breve, siamo nelle condizioni di guardare finalmente al futuro con maggiore fiducia e più sicurezza e con la consapevolezza di poter migliorare ulteriormente le condizioni di competitività del nostro sistema economico, proseguendo in un percorso che coniuga attenzione agli equilibri di bilancio e stimoli agli investimenti per una crescita strutturale e duratura. Il quadro è complessivamente diverso Il quadro è complessivamente diverso da quello dell'inizio della legislatura e ci ha visto duramente impegnati nel corso di questi anni. ultimi quattro anni, in particolare, la direzione impressa dai Governi è risultata da subito ben chiara e guidata dalla necessità di avviare un percorso di decisa ripresa economica e successivamente di alimentarla. Dopo un terribile tasso di riduzione del PIL, pari a meno 5,5 per cento nel 2009, e una seconda ricaduta di meno 2,8 per cento l'economia italiana nel 2014 ha finalmente mostrato un'inversione di tendenza e il quadro che abbiamo di fronte oggi, a tre anni di distanza, è ben diverso da quel momento, dell'inizio della legislatura. Due dati fondamentali ci confermano l'inversione di rotta. Il prodotto interno lordo, dopo un lungo periodo di difficoltà per il nostro Paese, si avvia verso un livello di crescita superiore alle attese nell'anno in corso, fino a raggiungere la soglia di 1,5 punti percentuali,

Il *deficit* pubblico - questo è il secondo elemento - è sotto controllo e si avvia verso un percorso che porterà al pareggio di bilancio nel 2020, mentre l'avanzo primario, che è previsto crescere nei prossimi anni, è tra i migliori tra i Paesi membri dell'Unione europea. Voglio dire che siffatti elementi si basano non su previsioni, ma sul fatto che in questi anni, ogni volta che è stato previsto un dato o un obiettivo, esso si è non solo confermato, ma ha anche superato le attese, a dimostrazione di una strategia che mette le basi su solide fondamenta. Negli ultimi mesi, poi, il ritmo della crescita si è accentuato in misura superiore alle attese e i benefici si riflettono anche sull'andamento del mercato del lavoro. Le politiche economiche, insieme alle riforme e alle diverse *policy* avviate negli ultimi anni, hanno restituito credibilità al Paese, in Europa e tra gli operatori economici e finanziari. E il decreto fiscale, collegato alla manovra di bilancio, si inserisce in questo contesto politico-economico, che va confermato, rafforzato e aiutato. Come anticipato, il provvedimento al nostro esame è parte di una manovra di bilancio complessiva. Esso contiene una serie di misure che contribuiscono, da un lato, alla copertura dei vari interventi previsti nella manovra tra questi cito la parziale sterilizzazione dell'IVA - e, dall'altro, a correggere l'andamento dei conti dell'anno in corso, con particolare riguardo ad alcune minori entrate, come quelle legate all'andamento della *voluntary disclosure bis* per meno 1,07 miliardi. Guardando agli effetti del complesso delle misure contenute nel provvedimento in esame e nel nostro disegno di legge di bilancio, si evidenzia che complessivamente gli impieghi proposti ammontano a 34,4 miliardi nel 2018, a 27,2 miliardi nel 2019

Il provvedimento, nel testo presentato al Senato, era articolato essenzialmente su quattro direttrici: in primo luogo, un pacchetto di misure fiscali, tra le quali si evidenziano l'estensione della definizione agevolata dei carichi, la riapertura della cosiddetta rottamazione dei ruoli, l'estensione del legalismo dello *split payment*, la sterilizzazione delle clausole IVA relative alle accise, l'estensione del credito d'imposta sulle campagne pubblicitarie a sostegno dei *media* e gli interventi fiscali in favore dei soggetti colpiti da quegli eccezionali e terribili eventi meteorologici dello scorso mese di settembre. La seconda direttrice è un insieme di interventi a sostegno delle imprese, quali il rifinanziamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, a cui si affiancano interventi per la trasparenza societaria finalizzati a disciplinare le scalate ostili, e misure per la difesa da minacce esterne di imprese strategiche per il Paese. Si modifica in questo modo la disciplina del *golden power*, con l'introduzione di soglie di possesso superate le quali l'acquirente è tenuto a dichiarare le sue intenzioni in termini di ulteriori acquisizioni di modifiche dei patti parasociali e degli organi di amministrazione. cito un insieme di misure di rifinanziamento legate al sistema generale della sicurezza, con il rifinanziamento delle missioni internazionali e la rideterminazione di piani di assunzione delle forze di polizia e del personale militare. è un articolato pacchetto di misure per affrontare diverse esigenze indifferibili. Voglio segnalare in questo ambito il rifinanziamento del fondo di occupazione e il monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica; la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana; la liquidazione della Croce Rossa Italiana e il finanziamento di obiettivi strategici di piano connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura e relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Questo è il testo iniziale. Nel corso dell'esame in sede referente, al di là anche degli argomenti contenuti nel testo originale del decreto o di alcuni direttamente o indirettamente a essi connessi, è stata affrontata in parte anche una serie di tematiche di interesse più o meno generale, alcune già emerse nel corso di precedenti provvedimenti (il decreto Mezzogiorno, la cosiddetta manovrina di giugno). In un clima di soddisfacente convergenza tra le forze di maggioranza, non meno che di sensibilità da parte delle forze di minoranza, è stato condotto un intenso e faticoso lavoro di costruzione, di mediazione che - grazie anche al costante e fattivo supporto del Governo - che ha mostrato un'ampia disponibilità al confronto, ha consentito di arrivare oggi in Assemblea con un testo condiviso. E per questo importante sforzo costruttivo voglio ringraziare tutte le forze politiche presenti in Commissione in questo Parlamento, il Governo e, in esso, in particolare, il vice ministro Morando. Durante i lavori in Commissione bilancio sono state apportate numerose e sostanziali modifiche di integrazione al testo, diverse delle quali provenienti anche dall'opposizione che, nel loro insieme, hanno confermato l'impianto generale del provvedimento e migliorato alcuni aspetti, ampliando significativamente i settori di intervento. Nel recepire, infatti, molte delle osservazioni emerse durante la fase istruttoria e consultiva congiunta per tutta la manovra di bilancio, alla fine sono state in parte chiarite, migliorate e integrate quelle previsioni che più delle altre davano adito a dubbi interpretativi, incertezza circa gli effetti concreti e perplessità riguardo il loro ambito applicativo. Mi riferisco, in particolare, alle misure fiscali contenute nella prima parte del provvedimento e alle misure sulle calamità naturali che hanno colpito varie zone del nostro Paese nel corso degli ultimi anni. Alla fase successiva della legge di bilancio 2018 è stata rinviata, anche in ragione dei tempi più ristretti a disposizione rispetto alla legge di bilancio, una serie di proposte (presentate anche in maniera *bipartisan*) che saranno approfondite ulteriormente nei prossimi giorni: il tema della previdenza, *in primis*, per il quale si è inteso rispettare il percorso di confronto avviato lunedì scorso e considerare che sulla materia è stato aperto un tavolo tecnico tra Governo e forze sociali; il tema del nuovo assetto delle agenzie fiscali, con particolare riguardo alla *governance* e all'inquadramento del personale; il tema della deducibilità, nell'ambito della più ampia tematica

la valorizzazione e il sostegno dell'attività dei *caregiver*. Sono temi centrali, non divisivi e maturi sul piano della priorità politica condivisa, ma non ancora definiti in parte sul piano legislativo, tanto da poter essere inseriti in questo provvedimento, ma certamente più realizzabili, anche per il tempo disponibile, nella seconda parte della manovra all'interno della legge di bilancio. Senza entrare nel dettaglio dell'articolato (per il quale si rinvia, per le parti non modificate, alla relazione che ho svolto in Commissione), mi soffermerò sinteticamente su otto principali modifiche approvate, cercando di aggregarle per grandi tematiche. In particolare, alle questioni fiscali, l'articolo 1, concernente l'estensione della definizione agevolata dei carichi, è stato oggetto di numerosi correttivi. Il termine per il pagamento delle rate, scadenti nei mesi di luglio e settembre 2017, relative alla cosiddetta definizione agevolata 2016, è stato posticipato al 7 dicembre 2017 (rispetto alla data inizialmente fissata al 30 novembre), che è l'unica data compatibile con gli equilibri di bilancio e la gestione delle entrate all'interno dell'anno 2017. Contemporaneamente si è provveduto a prevedere una proroga al mese di luglio 2018 del termine entro cui versare la rata di aprile 2018. È stata poi interamente riscritta la disciplina relativa alla cosiddetta rottamazione *bis* delle cartelle, avente a oggetto i carichi affidati agli agenti della riscossione, limitatamente dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, includendovi anche anche i debiti relativi a carichi affidati dal 2000 al 2016, per i quali non sia stata richiesta o non sia stata ammessa la rottamazione *ex* decreto-legge n. 193 del 2016. Ora riaprire questa opportunità per noi significa consentire ad altre aziende e a contribuenti di accedere alla possibilità fondamentale di chiudere pendenze con fisco e previdenza, che sono soltanto e soprattutto l'effetto del peso della crisi degli ultimi dieci anni, un peso che impedisce a quelle aziende la sopravvivenza e, se non essa, una piena ripartenza dell'attività economica. È stata poi incrementata di 8,9 milioni di euro nel 2018...

Grazie, Presidente. È stata incrementata di 9 milioni di euro circa nel 2018, 100 nel 2019 e 24 nel 2020 la dotazione finanziaria per far fronte a esigenze indifferibili del fondo per interventi strutturali di politica economica. Analogamente a quanto previsto per la definizione agevolata dei tributi locali riscossi tramite ruolo, sono stati allungati i termini per gli enti territoriali di deliberare la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento riferite alle entrate anche tributarie, notificate entro il 16 ottobre 2017, che è la data di emanazione del decreto in esame. Al fine poi di garantire l'integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali, è stato previsto che le funzioni e le attività di supporto e propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società a essi partecipate che spesso i Comuni esternalizzano, dandole in affidamento diretto a società di recupero e crediti, siano affidate a soggetti abilitati iscritti all'apposito albo. Tra le finalità a cui destinare in via esclusiva, a decorrere dal primo gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal Testo unico in materia edilizia, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2017, vengono inserite - questa è una novità - anche le spese di progettazione per le opere pubbliche. Infine, sempre sul tema fiscale, è stato rivisto lo spesometro ed è stata introdotta una serie di misure volte a semplificarne la disciplina, prevedendo in particolare, la non applicabilità delle sanzioni relativamente alle comunicazioni effettuate nel primo semestre 2017, data la natura sperimentale dei nuovi obblighi, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018; la possibilità che, al posto dei dati delle fatture emesse ricevute in riferimento alle operazioni rilevanti a fini IVA di importo inferiore a 300 euro, queste possano essere effettuate cumulativamente e possano essere trasmessi così i dati in un documento riepilogativo; luogo, l'esonero per le pubbliche amministrazioni dall'obbligo di trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali. All'articolo 4, poi, concernente gli incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari in materia di audiovisivo, è stata ampliata la platea dei beneficiari del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa e sulle emittenti radiotelevisive locali. Su questo tema sono state incluse, da una parte, le attività non commerciali degli enti non commerciali, mentre invece quelle commerciali erano state già introdotte. È un'apertura al tema del terzo settore, di tutto l'ambito del volontariato e dell'associazionismo. parte - anche questo è elemento di innovazione - gli investimenti possono riguardare a regime anche la stampa *online*, che costituisce ormai una parte rilevante del sistema della comunicazione e dell'informazione. Sempre in ordine al tema fiscale, faccio le ultime due segnalazioni. Siamo intervenuti in materia di decorrenza delle nuove disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore, stabilendo che per l'anno 2017 sono applicabili disposizioni agevolative vigenti anteriormente, quindi le nuove disposizioni a partire dal primo gennaio. E, quindi, sono pertanto deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore, nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque sino al massimo di 70.000 euro annui, le erogazioni fatte alle Onlus. a seguito della soppressione di Equitalia, la vigilanza, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, soprattutto per il rapporto con i contribuenti, viene svolta dal Ministero dell'economia e delle finanze anziché dall'Agenzia delle entrate, che ormai ingloba ciò che è

In questo ambito sono state approvate misure che contribuiscono a risolvere molte delle questioni ancora aperte relative alle calamità che hanno coinvolto L'Aquila, l'Emilia-Romagna, la Lombardia, il Veneto nel 2012 e le Regioni del Centro Italia nel 2016.

A queste misure, data la particolare gravità, si è aggiunto un contributo finanziario statale a favore della Regione Sardegna, a titolo di concorso alla concessione di indennizzi in favore delle aziende agropastorali che sono state danneggiate gravemente dagli eventi siccitosi registrati nel

è stato potenziato finanziariamente il settore dei confidi. L'incremento della dotazione del fondo di garanzia per le piccole e medie integrato dall'intervento di Cassa depositi e prestiti SpA. Si tratta di un'iniziativa che aumenta notevolmente le potenzialità finanziarie dei confidi e va nella direzione di sostenere, attraverso questo intervento, il mondo delle imprese. Ancora, la platea dei soggetti legittimati a partecipare al capitale viene allargato e si utilizzano le risorse, già attribuite al Piemonte, del fondo per lo sviluppo e la coesione per attribuire un contributo straordinario alla Regione di 35 milioni di euro per il 2017 e di 5 milioni per il 2018, al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto su gomma e ferro e far fronte così alla alla situazione finanziaria della società GTT SpA. Infine, con un intervento con un intervento dal sapore ambientale evidente, si incentivano gli investimenti in teleriscaldamento. Si tratta di una norma che intende estendere così le opportunità di produzione dei certificati bianchi e aumentarne la competitività in un mercato in cui solo pochi potevano produrli.

tra i quali ricordo l'adroterapia (una terapia importante sul piano della lotta ai tumori), viene previsto un intervento sulle neuroscienze e la neuroriabilitazione, sempre con il coinvolgimento di eccellenze di livello nazionale.

ampiamente allargato dal dibattito sviluppato in Commissione, che ha voluto integrare alcune opportunità, così da renderlo più completo dal punto di vista delle necessità nel territorio nazionale, con il determinante contributo di numerosi Gruppi politici di maggioranza e opposizione presenti in Parlamento. Voglio poi citare un intervento che riguarda gli studenti - ovvero le loro famiglie - nato per iniziativa parlamentare sul tema della detrazione degli affitti per gli studenti universitari. Questa può apparire una norma minore, mentre, in realtà consente di cambiare un'opportunità che, sino a questo momento, ha visto limitate le condizioni da parte delle famiglie i cui figli sono studenti universitari fuori sede. Oggi la norma vigente prevede la possibilità di detrarre la spesa dell'affitto per coloro che vivono oltre i 100 chilometri di distanza dalla sede universitaria, ma soltanto se si risiede in un'altra provincia. Con la modifica introdotta nel testo si estende la norma, riducendo a 50 chilometri la distanza per chi risiede in aree montane e disagiate - e ringrazio la proponente del testo e si elimina, attraverso l'intervento della Commissione, l'incomprensibile confine provinciale, considerando così universali i 100 chilometri di distanza in tutti gli altri casi. Si estende in questo modo la platea in maniera importante. Si tratta di un intervento

la questione concernente l'uscita dei minori di quattordici anni da scuola, emersa a seguito di una recente sentenza della Corte di cassazione. A tale riguardo si prevede che i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale

mediante una liberatoria che esonera il personale scolastico e gli enti stessi da ogni responsabilità connessa all'adempimento degli obblighi di vigilanza. La seconda questione di stretta attualità,

una pratica adottata sempre più frequentemente negli ultimi anni dagli operatori della telefonia mobile e della TV e che rischiava anche di diffondersi, con un meccanismo a tratti ingannevole nei confronti dei cittadini. Al riguardo si è introdotta una disposizione che, anche in linea con gli orientamenti successivi dell'*Authority*, prevede il ritorno della fatturazione su base mensile (o di multipli del mese) con la sola esclusione, nell'ambito della telefonia mobile, delle offerte promozionali temporanee. Per l'adeguamento alle nuove disposizioni da parte degli operatori si è previsto un periodo transitorio di quattro mesi. In questa norma - lo sottolineo, perché si tratta di un dato proposto da alcuni Gruppi - non sono stati inclusi i servizi pubblici, come acqua, gas e luce, perché servizi a consumo, il cui costo è indifferente al periodo di fatturazione. In questa normativa si è invece voluta integrare una regolamentazione riguardante i servizi forniti ai cittadini, introducendo l'obbligo di notificare al consumatore se il servizio offerto prevede l'arrivo della fibra sino all'abitazione o solamente sino alla centrale di prima distribuzione. Meno visibili, ma non meno attuali, sono due ulteriori interventi che voglio citare. Il primo è relativo alla sicurezza dei ponti sul Po, che richiede interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria necessari a garantire il transito dei mezzi tra le due sponde del fiume nelle strade statali - le uniche confermate e garantite sono quelle autostradali - in assenza dei quali il Paese rischia di rimanere diviso in due, in un punto nevralgico per le comunicazioni e l'economia del Paese. In secondo luogo, sono stanziate risorse in favore della Regione Lombardia

Sul piano ambientale voglio segnalare, oltre alla norma che permette di estendere la produzione di certificati bianchi, una norma di iniziativa parlamentare approvata dalla Commissione, che considero innovativa. A decorrere dal 2018 una quota pari al 5 per mille dell'imposta IRPEF potrà essere destinata anche a sostegno degli enti gestori delle aree protette. Si estende così, per la prima volta, all'ambito ambientale ciò che è stato previsto fino a questo momento per il sociale, prima, e per il settore culturale, poi, in questa legislatura, e che sta avendo un notevole e importante riscontro da parte dei cittadini. Ampliare la tematica sul tema ambientale consente di far diventare quella tematica non solo sensibile per i cittadini ma anche sostenibile per quelle sono le principali istituzioni nel settore ambientale del Paese. Cito come penultime le norme sul fronte dei trasporti. Qui i filoni sui quali abbiamo lavorato sono due: il tema della prevenzione dei fenomeni corruttivi e quello della sicurezza.

con un finanziamento di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2018: un intervento, come ho detto, previsto dal codice degli appalti, necessario per potenziare la prevenzione dei fenomeni corruttivi. Sul fronte della sicurezza segnalo due interventi: una misura sulla sicurezza del volo riferita alla condizione operativa del sistema dei controllori e l'introduzione - anche questa sollecitata in sede parlamentare e ampliata attraverso la collaborazione con il Governo - di una norma completa, e del relativo finanziamento, per allestire gli strumenti necessari a vigilare sulla sicurezza ferroviaria e marittima.

un intervento, anche di fronte ai recenti avvenimenti, che garantisca il mantenimento delle condizioni di continuità territoriale aerea con la Sardegna, che possono venir meno a seguito della cessione ad altri soggetti di Alitalia. con le convenzioni in essere, in caso di prosecuzione Alitalia abbia rinunciato ad alcune rotte, ed è importante che questo non avvenga se non in un contesto controllato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

a questa opportunità fino al limite del compimento dei trentacinque anni, ma i tempi più allungati della sottoscrizione della convenzione e dell'apertura del bando ci hanno ci hanno suggerito di estendere tale possibilità a chi aveva compiuto, alla data di approvazione della norma, il trentacinquesimo anno di età, mantenendo questo termine; quindi consentendo anche a chi ha superato quell'età - ma aveva i requisiti in quel momento - di poter accedere a «Resto al Sud». Abbiamo risolto in questa sede il tema dell'operatività rispetto al sostegno e all'attività tecnica di supporto di Invitalia. Cito poi altre due norme che mi sono particolarmente care per il dibattito e anche considerando che

che sono dovuti emigrare e che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa fuori dal nostro Paese e che dispongono di somme frutto di redditi regolarmente prodotti all'estero che possono essere utilizzate all'estero ma non in Italia. a queste somme, per cittadini italiani emigrati che hanno regolarmente prodotto all'estero il loro reddito, abbiamo ritenuto opportuno accettare una proposta che consente il rientro delle suddette per poter acquistare case nel nostro Paese, al fine di rientrare, come fanno tutti gli emigrati o la maggior parte degli emigrati italiani, mediante il versamento - del valore dell'attività e della giacenza al 31 dicembre 2016.

del nostro Paese, nelle pubbliche amministrazioni. Sono tre i territori che hanno subìto una diminuzione delle presenze di queste basi, e quindi il licenziamento di personale civile. Attraverso la norma consentiamo il finanziamento della cassa integrazione e avviamo il processo di ricollocazione

di un tema sensibile e sul quale pertanto occorre intervenire, anche perché diverse cause hanno generato il pagamento da parte dello Stato di risarcimenti ai militari che sono stati danneggiati o addirittura sono morti sono morti a causa di attività connesse all'attività militare. Pensiamo che prevenire tutto questo attraverso modalità di controllo ambientale e militare e una procedura di verifica costante del sistema di difesa - sulla quale so che esiste la disponibilità e l'accordo della Difesa

sul quale sono stato sollecitato e sul quale tutti i Gruppi politici hanno voluto un intervento. Lo tengo per ultimo perché è stato anche oggetto della parte finale, quella notturna, dei lavori di ieri.

Su questo voglio rendere merito al presidente della Commissione, senatore Tonini, perché questa norma era stata giustamente e correttamente espunta, per la legge di contabilità,

che comunque riteniamo possano essere regolamentati dal Ministero della giustizia. Era matura e necessaria l'estensione di tale principio agli altri professionisti. Per questo la norma introdotta, che inizialmente consentiva di evitare clausole vessatorie nei rapporti tra avvocati e sistema finanziario, cioè banche e assicurazioni, o grandi e medie imprese, viene estesa a tutti i professionisti, ordinistici e non. Inoltre, abbiamo inteso utile, e lo aggiungo, che oltre all'estensione agli altri professionisti, venisse inserito un richiamo che è di principio, nonostante esso sia vivo e insito nella nostra Costituzione, all'utilizzo dell'equo compenso da parte delle pubbliche amministrazioni. Non si di un richiamo alla qualità delle relazioni civili e al rispetto del lavoro quando esso viene reso, in particolare, all'interno del sistema pubblico del nostro Paese.

penso che il decreto fiscale collegato alla manovra concluda in quest'Aula il suo percorso e avvii il percorso della manovra più in generale. È un decreto che ha migliorato e incrementato gli obiettivi e i contenuti iniziali grazie ad un dibattito in Commissione fattivo e molto importante. Sono convinto che il Parlamento, con il suo dibattito, potrà potrà conformare che ciò che abbiamo integrato era atteso ed era utile. Sono convinto che il Parlamento, nel dibattere su questo provvedimento, potrà rilevare gli elementi positivi che aiutano il sistema economico, ma aiutano anche la coesione sociale del Paese.

perché il lavoro svolto era complesso e tenerlo nel giusto binario richiedeva attenzione e sostegno da parte di tutti e condivisione degli obiettivi. Questo è avvenuto e pertanto li ringrazio davvero tutti.

l'estensione della definizione agevolata dei carichi; la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari nei territori colpiti da calamità naturali; l'estensione dello *split payment* a tutte le società controllate dalla pubblica amministrazione; gli incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo; la parziale sterilizzazione dell'incremento delle aliquote IVA per il 2018; disposizioni urgenti in materia di missioni internazionali e disposizioni in materia di personale delle Forze armate; monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica e finanziamento del fondo occupazione; fondo di garanzia delle PMI; anticipazione delle risorse del fondo di solidarietà dell'Unione Europea; fondo imprese; procedura di cessione Alitalia; norme in materia di trasparenza societaria;

finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza; liberalizzazione in materia di *collecting* diritti d'autore; disposizioni finanziarie;

il decreto-legge è viziato senza dubbio da illegittimità costituzionale in quanto contenente disposizioni prive di collegamento formale con le tematiche richiamate dall'epigrafe del decreto e dallo stesso preambolo, l'eterogeneità delle materie in un decreto-legge determina un utilizzo improprio della decretazione d'urgenza e un depauperamento della competenza legislativa propria delle Camere, con conseguente svilimento del ruolo del Parlamento e l'affermazione di uno squilibrio dei poteri all'interno degli organi istituzionali a favore del Governo, più come un finanziamento a pioggia a fini politici che come interventi di carattere strutturale. Giova, altresì, ribadire che la *consuetudo contra legem* del legislatore di emanare decreti-legge in contrasto con sentenze della Corte indebolisce la credibilità degli organi legislativi, dei loro componenti e del valore del valore e della forza delle leggi e della Costituzione. L'inserimento di alcune disposizioni nel decreto-legge appare pretestuoso, posto che avrebbero potuto essere inserite nella prossima legge di bilancio *in itinere*, senza limitarne o inficiarne gli obiettivi che si prefiggono. Nello specifico del provvedimento gli articoli dall'uno al cinque, con riguardo all'eterogeneità, pur concernenti disposizioni riconducibili alla materia fiscale, affrontano questioni - come ho detto qualche attimo fa - tra loro diverse. L'articolo 1 reca l'estensione della definizione agevolata dei carichi, tema importante e sostenuto da Forza Italia tramite un proprio autonomo disegno di legge, assegnato alla 6a Commissione di cui non è mai iniziato l'esame. Esso ha subìto numerosi stravolgimenti che lo hanno reso farraginoso, di difficile comprensione e, molto probabilmente, non risolverà i problemi che coloro che sono in condizioni di grave o momentanea difficoltà finanziaria volevano fossero affrontati. Si tratta, al contrario, di una materia che necessitava un opportuno approfondimento e non dell'emanazione urgente di norme sicuramente inefficaci. L'articolo 3 estende il meccanismo dello *split payment* anche a enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, fondazioni partecipate e società quotate inserite nell'indice FTSE MIB. Questa ultima previsione finirà per togliere liquidità alle imprese, tagliando loro risorse, e sortirà l'obiettivo opposto a quelli di politica economica del Governo di rilanciare gli investimenti e la crescita; L'articolo 5 reca la parziale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA previsti per il 2018. Oltre ad essere sprovvista dei requisiti costituzionali essa è manifestamente illogica perché "sterilizza" 804 milioni di euro, lasciando altri 14.932 milioni di aumenti ancora pendenti sulla imposta sui consumi. "Sterilizza", inoltre, 304 milioni per il 2019, lasciando vigenti aumenti di IVA per 18.547 milioni di euro. L'articolo 8 reca un incremento, per l'anno 2017, del Fondo sociale per occupazione e formazione nella misura di 200 milioni di euro; la misura prosegue anche per gli anni successivi. Non si trova nemmeno in questa norma una adeguata giustificazione al suo inserimento in un provvedimento d' urgenza. L'articolo 11 reca un aumento al Fondo crescita sostenibile per il 2018 creato da un decreto-legge del 2012. Ora si crea, improvvisamente, una riserva di 300 milioni per tale Fondo senza avere chiaro se potrà essere utilizzata perché, oltretutto, l'eventuale utilizzo delle somme di tale Fondo, in soccorso di grandi imprese in difficoltà, deve passare il giudizio della Commissione europea per evitare l'eventuale apertura di procedure di infrazione per aiuti di Stato. L'articolo 12 reca il posticipo al 30 aprile 2018 del termine per il completamento delle procedure di cessione dei complessi aziendali di Alitalia. Anche per questo tema è singolare che si voglia trovare una soluzione, che certamente non sarà definitiva, in un provvedimento di necessità e urgenza. L'articolo 13 autorizza la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma, parte investimenti 2017-2021, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana. Anche questa norma, di preminente carattere ordinario, in quanto va a modificare il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, avrebbe potuto e dovuto trovare un'adeguata sede legislativa, perché non è certamente lo strumento del decreto-legge quello più adeguato a modificare la disciplina contenuta nel testo unico. Anche le disposizioni dell'articolo 14, che potrebbero essere definite gergalmente "chiudere le porte della stalla dopo che i buoi sono scappati", introduce modifiche al nostro ordinamento in materia di disciplina della cosiddetta *golden power* ovvero il potere di verifica pubblica sul controllo di aziende private. Norma che, anche laddove ritenute necessaria, non trova alcuna imminente giustificazione dell'urgenza ad esse assegnata. L'articolo 17 reca, ancora una volta, disposizioni per il finanziamento della bonifica e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera. Essendo un intervento più volte ripetuto e più volte non risolutivo, esso è per sua stessa natura non urgente. L'articolo 18 riguarda il finanziamento dei livelli di assistenza per un importo di 21,5 milioni, cioè per una somma che avrebbe potuto essere rinvenuta nell'ambito del bilancio dello Stato a legislazione vigente senza dovere adottare un apposito articolo L'articolo 19, che riguarda il recepimento di una direttiva europea in materia di diritto d'autore, viene inserita in questa sede, ma è evidente come vi fossero sedi più adeguate, quali ad esempio la legge europea. Una disposizione che, peraltro, andando a modificare il modello della gestione dei diritti d'autore (sinora monopolio della SIAE), risulta esso stessa una disposizione disposizione di carattere ordinamentale, totalmente inadeguata nella sede di un decreto-legge. La debolezza, a nostro parere, del provvedimento è nel proporre interventi legislativi che mirano a risolvere problematiche che avrebbero già dovuto trovare soluzione da tempo. In pratica, la decretazione d'urgenza sembra voler porre rimedio ad una mancanza di analisi preventiva ed accurata di un problema. L'assenza di verifica e di controllo di come una situazione di criticità evolve determina, infine, obbligatoriamente, la necessità da parte del Governo di dover intervenire nuovamente, improvvisamente ed urgentemente, per evitare che la situazione peggiori o continui a rappresentare un problema per il Paese. Tuttavia, affrontando una situazione in questo modo, difficilmente una situazione critica trova stabilità, potendo probabilmente degenerare in cronicità. In conclusione, la giustificazione dei requisiti costituzionali non si registra nemmeno nel complicato intrigo di commi, lettere e punti dell'articolo 20, che reca le disposizioni per l'utilizzo delle risorse e la copertura finanziaria delle norme inserite nel decreto-legge.

Siamo di fronte, signori colleghi e cittadini, alla degenerazione di un sistema parlamentare e c'è evidentemente uno squilibrio istituzionale fra il Parlamento e il Governo,

Gli articoli 13 e 14, ad esempio, sono stati inseriti nell'esame in Commissione e costituiscono un intero disegno di legge recante la riforma delle Agenzie fiscali, quindi stiamo parlando di una norma esattamente, perfettamente e strutturalmente ordinamentale.

Colleghi, la senatrice Stefani ha ragione, ve l'ho chiesto anche prima: per favore, un po' di rispetto per chi sta parlando. Mi scusi a nome di tutti. STEFANI *(LN-Aut)*. Grazie Presidente, ma non è cambiato niente. L'incostituzionalità di alcune norme è palese;

In questo caso, il personale si è ritrovato assunto dall'ente riscossione dell'Agenzia delle entrate senza avere nemmeno esperito un concorso pubblico, violando palesemente l'articolo 97 della Costituzione. Parliamo poi di un'altra materia che è veramente difficile e spinosa: lo *split payment*, lo *split payment*, che è già in entrato in vigore e che in questa norma viene ampliato ulteriormente. Crea un'evidente diseguaglianza e disomogeneità di trattamento tra i cittadini.

opera (clienti e professionisti) con le pubbliche amministrazioni e chi, invece, opera nel privato. Signori, è facile: nel privato si fa una compensazione dell'IVA e si hanno delle modalità con le quali si riesce a rientrare in qualche maniera e, invece, con questo sistema ci si trova con un problema di liquidità che deve essere anche affrontato.

che riprogramma i soldi stanziati per gli esodati riducendo il numero di richieste di accesso all'ottava salvaguardia, è in contrasto con i principi di diritto sociali

per l'ennesima volta si posticipa la fine dell'intervento dello Stato nella gestione di Alitalia attraverso la procedura di amministrazione straordinaria. Signori, l'articolo 41 riconosce la libertà dell'iniziativa economica Qui, invece, dal 2008 ad oggi lo Stato, riconoscendo questa condizione di crisi della società di bandiera, ha avuto un'ingerenza fortissima in numerosissime occasioni elargendo dal 2008 al 2014 una somma pari a 4,1 miliardi di euro, per non dire del resto. Siamo di fronte a un momento di grande crisi nazionale. sono state destinate per il risanamento di Alitalia, ma continuare a destinare ulteriori risorse pubbliche, distogliendole, tra l'altro, da altri interventi volti a far uscire il nostro Paese dalla crisi, crea sicuramente delle perplessità

Signora Presidente, intervengo sull'ultimo pezzo della relazione del senatore Lai, cioè sull'acquisizione, rispetto al testo iniziale, di un importantissimo... oggi siete indisciplinati. Cerchiamo di far parlare i colleghi. Se dovete allontanarvi dall'Aula, fatelo in silenzio. Aspettiamo un attimo, senatrice Parente, perché vedo che ci sono diversi senatori che stanno uscendo, così proviamo ad ascoltare.

La tutela del lavoro autonomo, compreso quello dei professionisti, è stata un crescendo in questa legislatura. Abbiamo approvato per la prima volta nella storia della Repubblica un disegno di legge che riguarda tutto tutto il lavoro autonomo, dai collaboratori ai professionisti, e abbiamo aumentato le tutele per questo mondo, l'intero mondo del lavoro autonomo. abbiamo condotto in questo Parlamento una battaglia, anche della maggioranza rispetto al Governo, per rendere stabile la copertura della cassa integrazione per le collaborazioni, la Dis-Coll. Oggi, nel decreto-legge fiscale, arriviamo all'equo compenso dei professionisti. Da mesi in Senato, nella Commissione lavoro, affrontiamo questo tema e io sono relatrice di un provvedimento al riguardo. Le norme che stiamo approvando oggi riguardano la necessità di un equo compenso per i professionisti, a cominciare dagli avvocati. Ricordava il senatore Lai che l'emendamento del relatore recepisce già una legge

riesco a capire come mai vi sia questa fibrillazione: c'è fermento, ma bisognerà smettere, per rispetto ai colleghi. Per favore, uscite dall'Aula se volete discutere tra voi.

PARENTE *(PD)*. Le norme che stiamo per approvare riguardano la necessità di un equo compenso per i professionisti, a cominciare dagli avvocati. L'altro ramo del Parlamento ha approvato una legge *ad* *hoc* per l'equo compenso degli avvocati e l'emendamento del relatore recepisce quel testo di legge.

è basata sul concetto di equo compenso rispetto a uno squilibrio contrattuale

è passata anche la richiesta, importante, di stabilire un principio nei confronti della pubblica amministrazione. Questo è importante soprattutto per i professionisti (dagli avvocati agli architetti e agli ingegneri),

aggiustare in questa norma, a cominciare dal riferimento più preciso a parametri rispetto ai quali si considera un equo compenso; questo potrà essere normato da decreti specifici dei Ministeri competenti. Noi che stiamo affrontando tali questioni da mesi nella Commissione lavoro abbiamo ascoltato i diversi mondi, dai rappresentanti degli ordini, ai professionisti non ordinisti; riceviamo moltissime lettere e siamo a conoscenza di tantissime esperienze,

ancora più specifico rispetto a questi temi. Noi abbiamo ritenuto che questa fosse una necessità anche nel decreto fiscale, perché abbiamo guardato soprattutto ai giovani professionisti, sia quelli iscritti agli ordini, sia quelli non ordinisti, e,

affrontare, oltre al riutilizzo dei fondi non spesi dell'APE sociale, anche il tema del prolungamento dell'APE sociale 2019 e personalmente ho presentato un emendamento alla legge di bilancio sulla questione dell'allargamento di tali misure a tutti i disoccupati, poi c'è il tema dei lavori gravosi, che sta affrontando il tavolo tra

fiscalità connessa alla vicenda dei terremoti. È un tema molto importante, sul quale noi abbiamo lavorato molto in questo fine di legislatura, e a partire dallo scorso anno. Purtroppo, come ho detto qualche istante fa, questo tema riguarda i terremoti, un fenomeno che coinvolge tutta la nostra penisola siamo resi conto di come, nel corso del tempo, questi provvedimenti vadano modulati in base a quello che poi scopriamo sul terreno. In particolare, mi riferisco alle

esiste un ovvio e purtroppo gravissimo danno strutturale e sociale prodotto dai vari sismi, ma poi si genera un cosiddetto danno indiretto,

si è verificato anche questo fenomeno e si è verificato con effetti molto pesanti. Quindi, anche città che non sono assolutamente coinvolte da

rimanesse agli atti e che ho già illustrato in Commissione e ringrazio il Vice Ministro, che ha posto molta attenzione sulla questione.

delle quattro Regioni, la percentuale delle attività che hanno messo a disposizione le loro strutture per quella che - ripeto - inizialmente abbiamo chiamato ospitalità

nella famosa soglia del 25 per cento di calo del fatturato non venissero ricompresi gli introiti dovuti alla ospitalità sociale. Poiché quelle strutture che,

senatore Puglia.

senatore Cioffi.

bisogna poi declinarlo, perché bisogna far sì che questi concetti trovino reale attuazione. Ribadisco che il problema non è reintrodurre il minimo tariffario, così come è previsto nel

sappiamo che esse sono soggette a gara, com'è giusto che sia e come è previsto anche dal codice dei contratti pubblici. Tali gare hanno prodotto affidamenti affidamenti con dei ribassi, com'è giusto che sia, ribassi che variano mediamente, secondo le statistiche che possiamo leggere, tra un valore massimo del 41 per cento e valori che stanno intorno al 26-27 sulle vecchie tariffe - che adesso sono «tabelle» perché abbiamo cambiato il modo di chiamarle - ci sono degli sconti che utilmente possono venire applicati. Introdurre il concetto di equo compenso - che poi sarà compito del Parlamento e del Governo declinare significa evitare quello che il Consiglio di Stato ha detto che si può fare, perché se la politica pensasse che tutto il sistema delle libere professioni si può reggere sul concetto che il compenso economico è scisso dalla corresponsione di un pagamento, allora saremmo ridotti male: vorrebbe dire che il

perché non è in questo modo che si risolvono i problemi, ma dobbiamo concentrarci sulle cose che abbiamo detto. Se chiediamo che tutto il sistema delle opere pubbliche

legali. Dobbiamo trovare un sistema, che contemperi l'esigenza di poter lavorare e di rendere una prestazione fatta bene alla pubblica amministrazione, con la necessità di lavorare per guadagnare e per vivere. Ciò significa non strapagare le professioni tecniche, un progetto o qualsiasi

tanti cittadini italiani provano a lavorare nella libera professione (e sono tanti i liberi professionisti nel nostro Paese) decidendo di stare Paese) decidendo di stare sul mercato - perché un libero professionista sta sul mercato tutti i giorni, per cercare di trovare un modo per vivere, ed è giusto che sia così perché ha scelto di stare sul libero mercato - non si può demolire tutto questo, in questo modo. Dunque mi auguro che il Governo ma probabilmente spetterà al prossimo Governo e al prossimo Parlamento - facendo sì che la dignità di tutti i professionisti in Italia sia rispettata, nell'ottica di fare bene il proprio mestiere e di rendere un servigio ben fatto alla pubblica amministrazione.

aiutare il lavoro e dare la possibilità alle famiglie di essere aiutate. In particolare,

richiesta è stata accolta - la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi, proprio a sostegno delle popolazioni residenti della ripresa delle attività produttive colpite dal sisma. È fondamentale che lo Stato in questi casi si faccia sentire in maniera robusta, che si faccia sentire sul fronte sociale.

misure in materia fiscale al fine di favorire la ripresa produttiva del settore turistico, che è fondamentale per quella zona, e poi, ovviamente, dei servizi connessi al turismo, pubblici esercizi e commercio. visto che parliamo di sistema fiscale, vige ormai da anni in Italia un qualcosa che a nostro avviso va assolutamente corretto: il cosiddetto acconto IRPEF, che si va versare nello stesso momento in cui si stanno versando le tasse dell'anno. Anzitutto, crediamo che, in maniera seppur

la cosiddetta mazzata. Ecco, crediamo che questo faccia male alle famiglie, alle imprese e all'economia del nostro Paese.

Già la spiegazione ci fa capire che è un sistema veramente complicato. Quindi, abbiamo chiesto una semplificazione,

hanno incendiato, la scorsa estate, il Sud Italia e, in queste settimane, il Nord Italia, prendiamo i soldi, le risorse finanziarie e umane e diamoli al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Chi sbaglia paga. Benissimo, ma anche lo Stato deve pagare nel momento in cui sbaglia. Noi riteniamo che sarebbe opportuno che lo Stato paghi nel momento in cui sbaglia e quindi, se una cartella esattoriale è stata notificata oltre la decorrenza del termine di decadenza o prescrizione, ancorché

concetto si applica al contribuente ma bisogna applicarlo anche per lo Stato, così vediamo se si lavora o non si lavora. Addirittura, poiché le cartelle esattoriali prescritte da oltre dieci anni che (nonostante questo)

Molto spesso ci riempiamo la bocca con il dire che l'Italia è un grande villaggio turistico e che l'Italia dovrebbe vivere soltanto di turismo. Sì va bene, questo è detto con la bocca, ma vogliamo fare degli atti concreti? Per

la seduta dell'Assemblea, a differenza di quanto era stato detto, sarà sospesa dalle ore 12,30 alle ore 16,30, in conformità a quanto stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, che ha affidato

Presidente, credo che il lavoro che deve fare il Governo, come quello che deve fare l'opposizione, in queste fasi dovrebbe essere improntato alla massima serietà e certamente sia la proposizione di questo decreto-legge fiscale come panacea di tutti i mali,

modalità che condividiamo. Bisogna essere molto precisi, non si possono fare elenchi come quelli che abbiamo appena sentito, andando a promettere rose e fiori, miele e latte che scenderanno dal cielo automaticamente. Quello che ci saremmo aspettati e che ci aspettiamo dal Governo, soprattutto in una fase conclusiva di legislatura come questa, in cui è evidente che molto, rispetto alle grandi prospettive di riforma che avevano caratterizzato l'inizio della legislatura, è mancato, è un'azione di pragmatismo. di pragmatismo. Non andrò a fare una disamina punto per punto, perché oggettivamente, come dicevo poc'anzi, gli elenchi "alla qualunque" non servono a nessuno, ma alcune considerazioni credo siano pertinenti e di merito.

Questo significa che nel momento in cui il legislatore - in questo caso mi riferisco direttamente al Governo, con i decreti-legge - entra in campo, lo fa senza aver pesato realmente il contenuto ed il merito di ciò che va a normare con legge e soprattutto non andando a fare delle

Mi stupisco molto nel rileggere ancora, in questo provvedimento, signora Presidente, di azioni emergenziali riguardo al terremoto. E non mi stupisco perché non conosco la situazione, anzi, la conosco molto bene; mi stupisco che, dopo un anno, qui dentro si sia ancora ad argomentare come emergenziale una situazione che, nei fatti, lo è ma che dopo un anno e qualche mese, rispetto ad agosto 2016,

delle strutture terremotate sono ancora a terra e le macerie neppure rimosse. Abbiamo scritto, signora Presidente, e abbiamo interloquito - ritengo in maniera utile - con il nuovo commissario alla ricostruzione, evidenziando circostanze che qui dentro sono ancora marginalmente toccate.

che ancora oggi in molti casi è oggetto di contenzioso con lo Stato, che non ripaga ai cittadini ciò che hanno fatto direttamente per trovare una soluzione abitativa, piuttosto che per risolvere direttamente la propria situazione di terremotati o, ancora peggio, penso a quella che è la situazione del mondo economico. Che per ricostruire queste città, questi paesi, ci vogliano anni, era noto fin dall'inizio; che per ricostruire il tessuto economico e produttivo ci vorranno molti anni è evidente. Come si può, allora, pensare di porre scadenze fiscali a distanza di qualche mese, a distanza di dodici mesi e poi essere qui oggi, con questo decreto-legge, a rinviare e spostare in là, di ancora sei mesi e un anno?

rabberciate e non capaci di dare ai nostri concittadini la certezza di uno Stato che non si ricorda della situazione solamente nella fase emergenziale, quando arriva una *troupe* televisiva, ma compie un'azione seria perché è giusto che sia fatta e non perché bisogna farla a favore di telecamera. Io sono stufo, signora Presidente, stufo di vedere le telecamere che girano in quei paesi e che inquadrano delle strette sezioni del paese trascurando la realtà che invece sta attorno, che è totalmente paralizzata. Lo abbiamo detto: era impossibile valutare il parametro economico degli incassi in funzione del breve periodo tra il settembre 2016 e il dicembre 2016, perché, paradossalmente, nel periodo corrispondente dell'anno precedente c'è stata una flessione mentre nel 2016, anche grazie alla solidarietà e all' aspetto emotivo, vi sono state vendite delle scorte dei magazzini crollati e di tutto ciò che poteva esserci in quelle zone, che falsano il dato di bilancio delle società. Ci troviamo, quindi, paradossalmente con società, artigiani e produttori terremotati che vengono esclusi dai benefici delle zone franche urbane perché il periodo considerato non mette in evidenza un calo di fatturato. Questo è falso. Non è così. Abbiamo allora insistito perché sia considerato un più ampio periodo e un più ampio segmento. Stesso discorso vale per gli aspetti contributivi. Si può pensare che, nel momento in cui qualcuno torna ad abitare in un *container*, lì si sia rimesso in moto un sistema produttivo, commerciale, industriale ed artigianale che consenta di riavere economia in autosussistenza? No. Lo dico al Governo: occorre seriamente una visione che vada ben oltre il quinquennio sulle esenzioni fiscali in queste zone e in queste aree.

«L'articolo 12 estende sino al 30 aprile 2018 il termine per l'espletamento delle procedure di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia in amministrazione straordinaria, che sono in corso di svolgimento. Conseguentemente anche il prestito statale oneroso di 600 milioni di euro, già disposto a favore di Alitalia, è integrato di ulteriori 300 milioni e la sua restituzione è prorogata fino al 30 settembre 2018, al fine di garantire la continuità del servizio (…)». Rinviare i problemi e non affrontarli non significa risolverli; significa distribuire e far pagare ai cittadini un ulteriore costo di una società che - lo abbiamo capito - nel tempo è stata cotta, ricotta e decotta, Presidente, su queste cose bisogna essere molto seri e determinati nel dare un segno al Paese che le politiche che vengono realizzate hanno lo scopo di risolvere i problemi, non di spostarli più in là.

bisogno di una grande riforma di responsabilità, che porti le nostre Regioni e i nostri concittadini a sapere che i loro soldi e le loro risorse sono amministrati dalle responsabilità più vicine, quindi dalle Regioni, non da un Ministero lontano che non fa altro che tagliare linearmente, senza andare a vedere il merito di chi sa ben spenderle o di chi le spreca. Bisogna dar corso velocemente a quella riforma o meglio, a una devoluzione di poteri che da sola può far risparmiare allo Stato

che circola sul *web* in cui si vede il Presidente della Repubblica che, guardando i terremotati, dice: «Non ci siamo dimenticati di voi, infatti, siamo qui a chiedervi di pagare le tasse». È il paradosso di un Paese che asseconda l'Unione europea,

nelle more dell'accredito dei contributi dell'Unione europea a carico del Fondo europeo di solidarietà, al fine di assicurare la tempestiva attivazione degli interventi a favore delle aree del Centro Italia colpite dal sisma». State parlando di «tempestività», quando da un anno le macerie sono ancora lì per terra; state parlando di un'Unione europea, a cui date continuamente il fianco, che neppure trasferisce i fondi e obbliga gli italiani a fare l'anticipazione sulle proprie risorse! No. Non siamo soddisfatti e non siamo contenti, soprattutto per la mancanza di concretezza in queste azioni. Il Paese ha bisogno di uno *choc* fiscale, della riduzione del carico fiscale sulle imprese.

Basta parlare di finanza; si torni a parlare di lavoro. Solo con il lavoro si crea ricchezza, solo con la ricchezza creata dal lavoro si può ridurre il debito pubblico e l'indebitamento degli italiani.

il decreto fiscale n. 148 del 16 ottobre 2017 in discussione ha il duplice compito di coprire i buchi di bilancio dello Stato 2017, determinati principalmente dal fallimento delle collaborazioni volontarie (meno 1.070 milioni di euro di entrate rispetto alle previsioni) e realizzare risorse per la legge di stabilità 2018. Il Governo fa cassa attraverso la riapertura dei termini per il pagamento agevolato dei carichi fiscali (30 giugno 2018 per 701 milioni), le liti fiscali pendenti (400 milioni), l'estensione dello *split payment* anche a tutte le società controllate dalla pubblica amministrazione (57,7 milioni), la proroga delle concessioni dei giochi (800 milioni, di cui 50 nel 2017). Il Governo procede alla riduzione delle risorse a disposizione dei Ministeri per un miliardo e 92 milioni. Le maggiori entrate così previste vengono utilizzate per coprire la sterilizzazione dell'aumento dell'aliquota IVA ridotta e delle accise sui prodotti petroliferi (840 milioni), per il finanziamento del fondo sociale per l'occupazione (200 milioni), per il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (300 milioni), il finanziamento di interventi sulla rete ferroviaria (420 milioni) e per le missioni internazionali (140 milioni). Il provvedimento rinvia alla legge di stabilità il macigno, che pesa sul bilancio dello Stato, rappresentato dalla clausola di salvaguardia dell'aumento delle aliquote IVA, che complessivamente pesano per 15.742 milioni, 14 dei quali sono a carico del bilancio 2018. Ovviamente questa clausola assorbe quasi tutte le risorse disponibili. Si fa per dire perché, in parte, provengono dalla magnanimità della Commissione europea che autorizza a fare ulteriore debito per 11,2 miliardi. Intanto, ad oggi, la Banca d'Italia ha comunicato che il debito pubblico ha raggiunto la quota di 2.283 miliardi. Siamo di fronte all'ennesimo provvedimento *omnibus*

All'ultimo momento in questo provvedimento sono stati inseriti numerosi emendamenti che, di fatto, lo stravolgono rispetto alla versione iniziale.

stato alcun dibattito, confronto e neanche la possibilità di apportare alcun contributo. Il provvedimento, inoltre, contiene norme per far fronte alla crisi sismica del 26 agosto 2016 e seguenti. ormai le norme che riguardano il terremoto sono distribuite in cinque provvedimenti. Altre norme sono contenute anche nella legge di stabilità. Siamo a sei provvedimenti. È possibile che ci vogliono sei decreti‑legge per affrontare una calamità come il terremoto? È possibile che non si possa adottare un provvedimento chiaro e comprensibile alle imprese, ai cittadini e ai professionisti? Ovviamente questa situazione, sulla quale mi voglio soffermare, ha determinato il fallimento dell'opera di ricostruzione. Nel provvedimento in esame noi avevamo proposto una serie di emendamenti suggeriti dai sindaci dei Comuni terremotati, che ovviamente avete ignorato. Intanto, bisogna chiarire un punto: in questo provvedimento non mettete soldi per il terremoto, ma vi limitate ad anticipare altri 300 milioni parte del miliardo gentilmente concesso dalla Comunità europea. Ad oggi le macerie sono quasi tutte lì, i camposanti sono ancora nella condizione in cui sono stati ridotti dalle scosse, gli interventi sulla viabilità sono interamente da realizzare (c'è voluto più di un anno per riaprire la Valnerina) e le casette sono ancora in alto mare. Erano state richieste dalle quattro Regioni colpite 3.702 casette, ma ne sono arrivate ad oggi (il dato è del 14 novembre) solo 1.228. Le Marche ne avevano richieste 1.843 e ne hanno avute 287. Ci sarà per i terremotati un altro inverno di precarietà. Il costo delle SAE (noi avevamo proposto di acquistare il patrimonio edilizio invenduto) è diventato incredibile, perché le urbanizzazioni costano cinque volte il prezzo al metro quadro della casetta. La ricostruzione leggera e pesante è ancora al punto di partenza e non siete riusciti neanche a trovare una soluzione praticabile per nonna Peppina, il cui caso ha esposto il nostro Paese al ridicolo agli occhi del mondo intero. Signor Vice Ministro, io l'avevo già spiegato in Assemblea, ma lei non l'ha voluto comprendere: per autorizzare la costruzione della casetta di nonna Peppina serve una deroga

Quindi voi la deroga la fate solo all'articolo 167 e non alle norme che possono consentire l'autorizzazione di questa costruzione. Abbiamo chiesto di spostare di qualche mese la scadenza per la compilazione delle schede AEDES, perché il 31 gennaio 2018 è un termine troppo vicino; ci sono infatti ancora migliaia di sopralluoghi da eseguire.

Vi abbiamo chiesto di trattare i marchigiani come avete fatto con gli abruzzesi (riduzione al 40 per cento degli importi da saldare), ma nulla di tutto questo Siete arrivati all'assurdo che un cittadino di un Comune terremotato, che ha avuta distrutta la casa e che si trova in zona rossa, non pagherà le rate dei mutui fino al 2020. Se uno però sta fuori dalla zona rossa, è costretto a ricominciare a pagare la rata la rata del mutuo, anche se obiettivamente non è ancora nelle condizioni di poterlo fare. Per quanto riguarda le scuole, tutte le gare che avete bandito sono andate deserte. Il bando prevedeva che le imprese che volevano partecipare alla gara per la costruzione e la riparazione degli immobili dovuto consegnare, insieme all'offerta, i progetti esecutivi, il che ha scoraggiato quasi tutte le imprese a farsi avanti (in pratica, pochissimi interventi sono partiti). Per le Marche si prevedevano 38 interventi, per un totale di 139 milioni, ma siamo al punto zero. Mi soffermo solo un attimo (perché il tempo scorre) sulla legalità. Voi avete un concetto della legalità sbalorditivo. Voi siete allergici alla legalità. La legalità la devono rispettare gli altri, mentre voi siete esonerati. Vi faccio un esempio concreto: la scuola di Amatrice

al quale è stata affidata la responsabilità di seguire queste 21 scuole, 18 da realizzare direttamente dal commissario e 3 costruite direttamente dai donatori. Questo giovane non ha le competenze per assumere un tale incarico, sia per il rilievo economico dell'opera, sia per il rilievo tecnico, perché si tratta di una struttura complessa. Il direttore dei lavori, signor Vice Ministro, è Fausto Cecchini, ingegnere *junior*: anche lui non ha il titolo di studio idoneo allo svolgimento di questo tipo di lavori. Il coordinatore della sicurezza è un altro architetto, Marco Pirri, proveniente dall'università di Roma; svolgeva un ruolo tecnico amministrativo e, anche lui *junior*, non ha le competenze. E la scuola va avanti nella più totale illegalità. Signora Presidente, concludo. Lascio da parte le polemiche tra il vecchio commissario Errani e Ceriscioli, ma non capisco se il Presidente della Regione parla o no con i commissari. I giornali di oggi riportano: «Ceriscioli scrive a De Micheli: "Procedure troppo complesse e farraginose per la ricostruzione"». Ancora: «Ritardi ingiustificati per le SAE. Serve semplificare l'*iter*». Ma tra il Presidente della Regione e il commissario è necessario scriversi o è meglio parlare? Non si è più efficaci se si prende il telefono e si spiegano le cose da fare? Ecco perché la ricostruzione è al palo: perché non avete saputo affrontare questa immane tragedia nei modi dovuti. *(Applausi

Signora Presidente, colleghi, saluto il vice ministro Morando in rappresentanza del Governo. Ringrazio il relatore

ringrazio anche il Presidente della Commissione bilancio. In sostituzione di un collega ho potuto condividere questa esperienza e trovo che, alla conclusione di queste giornate impegnative,

su moltissimi emendamenti vi è stata una convergenza che oggi non respiro. Sembra quasi che dalle 3 di questa notte alle 11 di questa mattina sia passato un abisso. Io non sono d'accordo, perché questi sono luoghi importanti; sono luoghi in cui il lavoro che abbiamo fatto nei giorni precedenti dovrebbe essere riportato con le adeguate lealtà e serenità. La verità è che abbiamo condiviso molte cose e che, anzi, su molte questioni la maggioranza ha fatto un passo indietro per poter dare ai colleghi dell'opposizione uno spazio d'azione. Questi sono i fatti. Ora, entriamo nel merito. Il decreto fiscale si occupa di molte, molte questioni e se ne occupa abbastanza bene. Se su qualcosa dovessimo ravvisare un'imperfezione, c'è il tempo - e questo il Vice Ministro l'ha detto più volte - di intervenire in legge di bilancio (iniziamo subito) per, eventualmente, aggiustare il tiro di qualche norma: tiro di qualche norma: penso alle zone franche per le aree terremotate o alle agenzie fiscali o ad altri argomenti che, proprio per la complessità e la durezza del confronto, hanno bisogno magari di qualche giorno in più. E lo faremo; lo abbiamo detto e lo facciamo.

Penso all'ampliamento della possibilità della rottamazione delle cartelle, alla neutralizzazione dell'aumento dell'IVA, all'incremento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, alle misure di sostegno alle imprese in crisi,

dove, per anni e anni, la normativa si è dovuta aggiustare. Mi stupiscono alcuni giudizi sommari, soprattutto degli esponenti del centro-destra

che invece questo Governo ha realizzato in automatico già con strumenti precedenti a questo, gli abruzzesi dovettero scendere in piazza, prendendosi anche le manganellate. Adesso, trasformare questo evento in una vicenda mitica si scontra con la realtà. Il problema fu che la sospensione delle tasse all'epoca e la restituzione parziale, che naturalmente aveva avvantaggiato i cittadini che ne avevano usufruito,

quindi evidente che c'è un percorso di modifica dello Stato, non delle maggioranze, nell'approccio a queste vicende, anche perché sul terremoto del 2009 è intervenuta l'Unione europea

terremotata la richiesta di restituzione di somme molto cospicue. Con il sottosegretario Gozi stiamo ora portando avanti una difficilissima mediazione affinché queste somme non debbano essere restituite.

avere una visione organica di terremoti che sono tutti diversi. In questa legislatura abbiamo affrontato il 2009, quando rimanemmo senza soldi e il Governo dovette mettere nel primo provvedimento il decreto sugli enti locali, 1,4 miliardi; il

problemi. Intanto, si parla di edilizia pubblica. Tutti sanno che per me è una fissazione, anche memore dell'esperienza. Con le regole normali (che ovviamente vanno salvaguardate, perché sono garanzia di efficienza, ma anche di legalità e rigore amministrativo) in stato di emergenza e anche nel *post* emergenza non si riesce ad appaltare.

paradossalmente, va più lenta di quella privata: nell'edilizia privata c'è l'immediata concessione del contributo, mentre in quella pubblica l'ente pubblico è tenuto a una complessa procedura.

che, specie nelle aree terremotate del Centro Italia (che sono tutte sottoposte a vincolo paesaggistico e alla normativa sui parchi,

importanti per il Centro Italia, oltre a quelli che ho citato. Penso alle proroghe dei contributi e al SIA aree sisma, che finalmente viene ai finanziamenti ai Comuni delle zone sismiche per i progetti della messa in sicurezza. Sembra niente, ma è tantissimo per chi ha vissuto quell'esperienza. Il Comune non ha i soldi per fare il progetto

l'impresa può restituire successivamente le somme, senza caricare sullo Stato il mancato rientro delle somme stesse. Il Governo, attraverso i provvedimenti (quindi lo Stato), si fa carico del tasso di interesse, che viene sostanzialmente annullato.

quando ha voluto dare subito la risposta con la zona franca. Avevo qualche perplessità, perché una zona franca può funzionare, in un'area terremotata, in un momento successivo alla prima fase dell'emergenza.

di entrate, ma addirittura alcune hanno registrato un picco: penso a quelle attività commerciali, che magari hanno dovuto sostenere l'emergenza, nel campo della panificazione o del commercio

Si interviene poi con la norma sulle procedure per l'edilizia scolastica e sulla possibilità per i Comuni dell'Aquila, che già lo ha fatto - di avviare un'azione per supportare la ricostruzione, con un'opera infrastrutturale di sottoservizi. Si

al terremoto, dipendenti a tempo indeterminato, vincitori di concorso indetto dal Ministero, che però non hanno un'allocazione stabile, ovvero sono prestati ai Comuni

debba essere affrontato, prevedevo la possibilità di protocolli di intesa con i Ministeri e gli enti locali, affinché si definissero delle postazioni, con una sorta di prenotazione,

perché, non sapendolo, cercano di trovare altre strade per avere una sede stabile e non rischiare di finire magari in una lista di mobilità. È un tema tutto tecnico e organizzativo, ma

cui, paradossalmente, quelli che sono nel susseguirsi della graduatoria vengono chiamati dai Ministeri e assunti, giustamente, a tempo indeterminato. Quindi, chi lo ha vinto, ha questa strana collocazione e chi non lo ha vinto direttamente, ma è comunque idoneo e in qualche modo abilitato, magari trova immediatamente una collocazione. Mi scuso se mi ci sono soffermata particolarmente, ma è un tema che sta determinando parecchie fibrillazioni nel funzionamento degli uffici e non vorrei che questo rallentasse il tiraggio della ricostruzione. Altro tema introdotto con l'emendamento del relatore

un qualche correttivo che, nella nottata dei lavori in Commissione, non è stato possibile apportare per la celerità e per la novità

si diano risposte importanti e adeguate, non perfette, perché non c'è perfezione in questo campo: non ci sono manuali né del buon terremotato né del buon amministratore che deve gestire il terremoto;

viene meno ogni sicurezza: perdere la casa, il lavoro, e magari qualche anima della tua famiglia ti porta in una condizione di totale insicurezza.

è in atto ancora adesso il tentativo pervicace di propinarci un emendamento in materia di servizi segreti, di sicurezza, sicurezza, in particolare la creazione di una fondazione di diritto privato a tutela della nostra sicurezza cibernetica. È un tentativo pervicace che ha avuto modalità e finalità nell'utilizzo di uno strumento opache e sbagliate. vicenda non si è ancora conclusa. Si tratta di un emendamento che è stato presentato in prima battuta al disegno di legge di bilancio, poi dichiarato inammissibile dal Presidente della Commissione bilancio. Una volta sparito, diventato fantasma questo emendamento, ce lo siamo ritrovato all'interno del disegno di legge fiscale. Sembra sia stato dichiarato ammissibile e poi, nella seduta notturna di ieri, nonostante messaggi di agenzia parlassero di un emendamento approvato, veniva ritirato dal Governo e ci viene ora annunciato che questo testo, che prevede la creazione di una fondazione di diritto privato in materia di servizi di *intelligence*, ricomparirà o al momento del voto di fiducia che verrà posto o, più probabilmente, durante la discussione della legge di bilancio. Si tratta di un tentativo pervicace, fino ad ora abortito, che va peraltro segnalato per motivi di carattere squisitamente istituzionale. Non si tratta certamente di un attacco ai servizi segreti, che anzi intendiamo tutelare, non si tratta di una sottovalutazione del livello di protezione cibernetica e della sicurezza informatica nazionali, che anzi vogliamo tutelare nella maniera più assoluta, non si tratta - lo dico pur da una posizione di opposizione - di un attacco al Governo, bensì di una richiesta di trasparenza totale, di una richiesta di rispetto delle istituzioni che viene rivolta in questo momento al Governo. Questo emendamento riprodotto, quasi fantasma, presentato al disegno di legge di bilancio e ripresentato per il decreto fiscale, fa riferimento alla possibilità che il Presidente del Consiglio dei ministri, ma in particolare il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, il DIS, presieduto dal prefetto Pansa in questo momento, possa costituire anche per la promozione di mirate attività di ricerca, una fondazione di diritto privato. Questa è una cosa strabiliante. Io ero venuto personalmente a conoscenza di questa vicenda nella giornata di lunedì. Non volevo credere a quello che mi veniva detto. Ho chiesto, fuori dall'attività del Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, e quindi ne posso parlare, chi fosse a conoscenza di questa vicenda. I membri del Comitato non sapevano niente. Abbiamo cercato di capire qualcosa ma neanche i Capigruppo di Camera e Senato di tutti i Gruppi sapevamo

se andiamo ad analizzare l'emendamento che è stato proposto per il disegno di legge di bilancio e pervicacemente riproposto per il disegno di legge fiscale, rimaniamo ancora più perplessi perché non vengono descritte le finalità di questa fondazione di diritto privato. Si parla anche della promozione di mirate attività di ricerca e non si sa quali siano ma soprattutto quell'«anche» ci desta preoccupazione. A che cosa fa riferimento e perché i soggetti privati devono essere chiamati ad intervenire direttamente nelle attività della

con gli istituti di ricerca attraverso convenzioni regolarmente previste dalla legge, che vanno comunicate al Copasir e che hanno tutta una loro procedura istituzionale corretta in modo tale che venga sempre garantito il massimo della trasparenza. Tra l'altro, devo dire che il fatto che il prefetto dirigente in questo momento del DIS venga audito e non racconti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di questa vicenda è già di per sé una questione che desta molte, molte perplessità. Il DIS, infatti ha moltissimi compiti. Basta scorrere rapidamente

la n. 124 del 2007, per renderci conto di come i poteri del DIS siano amplissimi. Facciano riferimento sempre alla Presidenza del Consiglio ma da nessuna parte, né per la parte che concerne i poteri e le competenze del DIS, né in altre parti, si parla di fondazioni di diritto privato, di soggetti privati se non in una maniera e in una misura istituzionale molto corretta. Infatti, dopo aver parlato, all'articolo 8 di questa legge, della esclusività delle funzioni attribuite al DIS, al servizio segreto esterno e al servizio segreto interno, cioè AISI e AISE, per quanto riguarda la materia e le funzioni dell'*intelligence*, si dice all'articolo 11 che possono essere stipulate convenzioni con soggetti e amministratori pubblici e privati, nonché con l'università e con gli enti di ricerca secondo l'ottica di tutela e di protezione anche, se non soprattutto, cibernetica e informatica. a seguito di queste norme, è stato fatto ampiamente ricorso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai sottoposti DIS, AISE e AISI, a convenzioni con le nostre università a decine, proprio per sottolineare ed ampliare anche l'attività di ricerca in materia di sicurezza informatica e cibernetica. Di fronte, quindi, ad un panorama normativo e di fatto di *intelligence* chiarissimo che funziona, che fino a questo momento non ha creato perplessità, ci troviamo di fronte ad un un emendamento di questo tipo, sul quale tra l'altro anche nella seduta di ieri sera il Gruppo Articolo 1 è intervenuto per chiederne la soppressione *in parte qua*, attraverso l'emendamento proposto dalla senatrice Ricchiuti, sottoscritto anche da me e dalla senatrice Lo Moro, proprio perché una situazione di questo tipo non può essere accettata (in conclusione dirò qual è il rischio che corriamo). Questo della fondazione di diritto privato - ripeto - è uno strumento sbagliato: quando abbiamo approvato nel 2007 questa legge, abbiamo preteso, voluto, valutato e votato per il massimo della trasparenza dei nostri servizi di sicurezza proprio per evitare zone grigie, opache, commistioni. Volevamo che tutto fosse pubblico, che tutto percorresse una strada chiara ed istituzionale e volevamo evitare norme di questo tipo che non si sa dove nascono e non si sa dove vanno a parare. Oltre a questo, ci sono delle modalità opache, perché non capisco per quale motivo i Capigruppo di Camera e Senato non fossero stati informati di una norma così rilevante che modifica l'impianto istituzionale della nostra *intelligence* e non si capisce per quale motivo - ci diranno poi corrisponde a verità - il capo del DIS contatti i vertici della Commissione bilancio del Senato per parlare direttamente di questa vicenda (è assolutamente al di fuori di ogni regola, quindi vorremmo anche capire che cosa, perché e come è successo su questa materia) e non si capisce che cosa vogliono con la creazione di questo fondo, senza appunto informare non forse vincolativamente, ma doverosamente il Comitato parlamentare e senza informare preventivamente le forze politiche che devono votarlo in Parlamento.

con quali finalità, con quali scopi? Mi rivolgo al Governo, perché siamo in grado di intervenire e di bloccare questa situazione, ma sarà da capire se questa che io definisco una "deviazione istituzionale" troverà gambe per andare avanti o verrà bloccata definitivamente in quest'Aula del Senato.

qualche decina di milioni in alcune parti, di qualche centinaia di milioni in altre, ma qui c'è un emendamento da 11 miliardi che è passato senza grande clamore, si tratta

ha comportato ricavi per 370 milioni, un margine operativo lordo tra i 160 e i 170 milioni e addirittura un utile un utile superiore ai 100 milioni. Questo, moltiplicato per i trent'anni per i quali vi è questo regalo, comporta undici miliardi (più uno per i tre anni già passati senza nessuna gara) di ricavi; cinque miliardi, più più mezzo, per quanto riguarda il margine operativo lordo e, addirittura, considerando solo l'utile, sono comunque due miliardi e mezzo. Questo a fronte di che cosa? Del versamento di settanta milioni per sette anni, cioè di mezzo miliardo. mezzo miliardo - in futuro, non subito - e, in cambio, dà via libera a cinque miliardi e mezzo che starebbero molto meglio nelle casse dello Stato, per le tante necessità che lo Stato ha, piuttosto che in una in una nuova municipalizzata. Io avevo sentito dire che questo Governo e quello precedente volevano ridurre le municipalizzate. Magari, invece, si massacrano municipalizzate, talora anche utili (non tutte sono inutili, infatti), da qualche decina di migliaia di euro,

settembre del 2011 aveva attivato le procedure per la concessione. Perché è buona norma attivare le norme per una gara dopo la concessione; non quando la concessione è ampiamente scaduta, come l'attuale Governo sta facendo per la Torino-Piacenza, ma prima. E il ministro Matteoli lo fece quasi tre anni prima della scadenza della concessione.

anni. Da lì potevano esserci le offerte al ribasso di coloro che partecipavano alla gara. Qui, invece, si è partiti dalla base e alla base si resta. Dunque, è un regalo enorme. Ci sono delle omissioni in quanto in questo emendamento non c'è alcuna delle condizioni né i vincoli previsti, invece, nell'appalto indetto dal Governo Berlusconi nel 2011. Qui non si parla di investimenti. Una riduzione tariffaria o, perlomeno, un contenimento degli aumenti non sono menzionati. Praticamente, una cosa che doveva essere fatta a gara, a competizione, è data in regalo per trentatré anni. Ora, io chiedo al Governo di avere il

Noi non capiamo. Ogni spiegazione che mi viene in mente è maliziosa, per cui non ne faccio alcuna. Chiedo al Governo che, anziché dare spiegazioni, non includa tale misura nel maxiemendamento. Queste cose si potranno fare in seguito. Se è nella convenienza dei cittadini, lo si potrà fare. Ma io ritengo che non sia convenienza dei cittadini fare di tutto per azzerare una misura che lo stesso Governo, da legislatore, ha inserito, cioè il divieto di proroga delle concessioni autostradali,

percentuali di partecipazione all'azionariato dell'autostrada siano rese pubbliche, possono chiedere il prezzo che vogliono. Quindi, altro regalo indebito. Il tutto giustificato con un vago rilancio degli investimenti. Le norme europee, il buonsenso e l'obbligo per i Comuni, per esempio, vogliono che i risparmi si ottengano facendo le gare, non i regali: c'è una bella differenza. Qui invece si è scelto di fare il regalo, lo

In quella Regione si passa da incarichi di dirigenza di uno dei due partiti indicati (il Partito Democratico e La Südtiroler Volkspartei) a una presidenza e una megadirigenza di quest'autostrada e dall'una all'altra. È sostanzialmente la stessa cosa. Qui si voleva abolire mezza Costituzione per risparmiare 50 milioni di euro all'anno e poi si regalano 5 miliardi e mezzo. Complimenti: chiedo al Governo di avere il pudore - ripeto - di non includere quest'emendamento nel maxiemendamento: sarebbe una vergogna e uno schiaffo agli italiani, nonché alle imprese che vorrebbero essere rese competitive. Ricordo che non siamo più - e non lo siamo mai stati - nei piani quinquennali dell'Unione Sovietica; qui siamo invece nei piani quinquennali - anzi, trentatrennali - di concessioni regalate, in attesa di fare altri regali ad altri concessionari, di cui leggiamo sui giornali.

il provvedimento che ci accingiamo ad approvare si compone di luci ed ombre. Riflette, in estrema sintesi, l'atteggiamento della maggioranza che sostiene questo Esecutivo e, ancora di più, lo stato d'animo e gli umori del principale azionista di questa maggioranza e di quella precedente.

Nel testo, alla fine, si è inserito un po' di tutto, compresa la norma che definisce i nuovi termini temporali degli incarichi di vertice delle Forze armate: l'ennesimo provvedimento *omnibus*. Altra nota dolente, che purtroppo torna a farsi sentire in questo ramo del Parlamento, è la tempistica data al dibattito. Mi riferisco, ad esempio, agli emendamenti del Governo legati agli eventi sismici,

ovvero con un risarcimento economico. Il Governo, dopo le polemiche politiche e delle associazioni in seguito al primo caso a Torino, che tutti conosciamo, ha deciso di intervenire per modificare la recente riforma al procedimento penale. Il risultato non è certo frutto di un'attenta riflessione dell'Esecutivo o di qualche suo egregio componente, ma della battaglia portata avanti dalle associazioni e da alcune di noi, che con forza hanno denunciato la gravità tante ombre e poche luci in questo provvedimento, dal quale ci si aspettava qualcosa in più: da un lato, ad esempio, sono certamente apprezzabili le misure in materia di *split payment*; dall'altro, suscitano perplessità le disposizioni in materia di definizione agevolata di cui all'articolo 1, che di fatto rischiano di dare luogo a una forma di condono reiterato. disposizioni che vanno incontro ad esigenze che definirei elettorali e che rischiano di configurarsi come un ulteriore incentivo a comportamenti scorretti nei confronti del fisco, come in particolare l'evasione da riscossione, peraltro già in aumento, con conseguenze fortemente negative sulla tenuta del sistema fiscale nel suo complesso.

Con questo emendamento si fa riferimento a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate. È una modifica importante che va nella direzione giusta e permette agli studenti di quelle zone di godere delle detrazioni

e questa forma di detrazione per chi studia e raggiunge con difficoltà scuole e atenei possano diventare strutturali ed essere di supporto alle famiglie che vivono in territori montani e in zone disagiate, con difficoltà e costi maggiori e diverse possibilità di accedere allo studio.

Siamo al secondo anno successivo alla soppressione della legge di stabilità che, come sappiamo, era stata lungamente tacciata di essere diventata un contenitore, un carrozzone circense di norme dal contenuto più disparato che ben poco avevano a che vedere con la materia di bilancio in senso stretto. Adesso che sono intervenute parecchie restrizioni su questo fronte, ho la sensazione che il metodo che il metodo equivalente di norme *omnibus* sia stato contagiato dal cosiddetto decreto-legge fiscale, tant'è che il provvedimento odierno contiene, in realtà, solo quattro articoli di natura strettamente fiscale (la rottamazione delle cartelle *bis*, l'estensione dello *split payament*, la sterilizzazione dell'aumento dell'IVA e la sospensione dei tributi per i territori colpiti da calamità naturali). Tutto il resto è veramente opinabile che possa ricondursi alla materia fiscale. Tuttavia, nello spirito di collaborazione e nel solco della ricerca del miglioramento del testo, avevamo presentato in Commissione dei buoni emendamenti che sono stati irrimediabilmente respinti. Mi riferisco, per esempio, alle disposizioni per lo sviluppo del settore librario nei Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti. Ci lamentiamo del fatto che gli italiani leggano poco, che investano poco in cultura e quindi sosteniamo che sono necessarie le misure incentivanti. Ma gli aiuti alle piccole librerie e storiche dei piccoli Comuni sono caduti nel vuoto. Ho presentato emendamenti riguardanti gli investimenti sui sistemi di trasporto intelligenti, fondati sull'interazione tra informatica, telecomunicazioni e multimedialità, che consentono di affrontare in modo innovativo i problemi della mobilità pubblica, collettiva e privata, sviluppando in modo organico e funzionale soluzioni improntate su sicurezza, efficienza, efficacia, economicità nel rispetto dell'ambiente. Ma anche queste proposte sono state respinte. Mi riferisco inoltre ad alcuni emendamenti di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di personale delle agenzie fiscali. Ebbene, neppure in questo caso ci è stato consentito di poter dare un contributo migliorativo, stanti le raffiche montanti di un voto di fiducia sempre più probabile. Quindi con rammarico dobbiamo constatare ancora una volta il ricorso del Governo allo strumento della decretazione d'urgenza per portare in Parlamento un provvedimento che, come del resto conferma la migliore tradizione di sinistra in voga in questi ultimi anni di legislatura, pecca nella forma e nei modi, rappresentando un ulteriore esempio di peggioramento della qualità della legislazione. Un provvedimento che si presenta come collegato alla legge di bilancio, di cui cogliamo carenze e inadeguatezze sul fronte dello sviluppo e della crescita. Manca una prospettiva concreta e credibile, manca una strategia efficace, manca una visione unitaria di proiezione in un futuro che pure deve essere preso in considerazione, che merita attenzione e disponibilità di intelligenza e di una *governance* credibile. O, per meglio dire, qui l'unica proiezione sembra essere sempre e solo quella elettorale. Proprio perché ci avviciniamo a grandi passi alla fine della XVII legislatura, temiamo che il Governo voglia utilizzare gli ultimi atti più per compiacere una parte di elettori cui si rivolge per tentare di risalire la china che per il perseguimento del bene complessivo del Paese. Quello che balza agli occhi in maniera eclatante è che nulla di veramente serio viene fatto per ridurre la pressione fiscale; anzi, possiamo dire che le disposizioni sullo *split payment* rischiano di tramutarsi in una tassa vera propria sulla liquidità per le imprese e i professionisti. E ancora sul Sud riscontriamo carenze di attenzione. Lo abbiamo detto tante volte e lo ribadiamo: il Mezzogiorno ha bisogno di interventi risolutivi, dal credito di imposta alla fiscalità di vantaggio, e non ha bisogno di qualche *spot* e di qualche misura cosiddetta *light* (leggera). Ancora una volta una beffa conclamata, che certamente amplifica il grado di inaffidabilità e inadeguatezza di questo Governo. Ci sarebbero altre ragioni di disapprovazione da elencare in merito a questo provvedimento, ma quelle appena enunciate costituiscono, a mio modo di vedere, un estratto sufficiente per manifestare tutto il nostro dissenso a questo provvedimento di conversione, che ancora una volta, nel merito come nel metodo, prova le carenze di un Governo che è ormai visibilmente proiettato in campagna elettorale e che arranca in cerca di consensi spiccioli, prestandosi a operazioni di piccolo cabotaggio, buone per accontentare qualcuno, ma che a guardar bene mancano di respiro e di visione e poco sono improntate ai principi di buona amministrazione.

capire che ci è d'obbligo osservare i fenomeni e attivare strategie precise. In Italia abbiamo un immesso sul mercato di circa 2,1 milioni di tonnellate di plastiche; ne raccogliamo 900.000 tonnellate e ne mandiamo al riciclo soltanto 540.000. C'è quindi un riciclato pari ad un quarto di quello che è immesso al consumo (questi sono dati di Assorimap dell'anno scorso). Perché succede questo? Eppure in Italia abbiamo delle tecnologie e degli impianti che ci rendono *leader* nel settore, ma, senza un sistema adeguato di valorizzazione di questa filiera, avviene che, così come i cervelli, si verifica una continua fuga di aziende verso Paesi che, a differenza nostra, attuano politiche economiche a vantaggio di chi veramente attua politiche di economia circolare. Circa il 50 per cento delle plastiche raccolte finisce in inceneritori o discariche; recentemente più in discarica che in inceneritore, perché gli inceneritori sono intasati. Il Plasmix, che è la parte meno nobile delle plastiche, fatto al netto delle PET e del polietilene (sono le cosiddette plastiche miste), sta avendo un aumento di produzione, perché c'è una maggiore richiesta di prodotti monouso e soprattutto di *packaging* finalizzati a un miglior mantenimento dei prodotti alimentari. Questi prodotti in Plasmix sembrano difficilmente riciclabili, ma non è vero. Sono, infatti, diversi decenni che la ricerca ha permesso di trasformare anche questi residui plastici in materia prima-seconda;

urbani, banchi di scuola, pannelli fonoassorbenti e tanto altro ancora. Ma è una filiera che non viene sostenuta e incentivata. Questi rifiuti, quindi, cercano un altro tipo di soluzione e finiscono negli inceneritori; questi, non potendoli ricevere,

negli ultimi anni sono centinaia gli incendi che avvengono in questi siti di trasferenza. C'è, quindi, una difficoltà a smaltire una materia che potrebbe entrare in una filiera economica importante. C'è qualcuno che, invece di proporre di fare veramente economia circolare e di fare nuova materia prima-seconda, propone nuovi inceneritori. Vi ho parlato solo di economia; chiaramente non ho neanche voluto sollecitare la vostra immaginazione sulle isole di plastica negli oceani e sul fatto, ormai accertato, che queste microplastiche sono entrate nella filiera alimentare.

che ha recentemente registrato un ottimo consenso e un apprezzamento proprio da Assorimap con un comunicato stampa dell'8 novembre scorso, denominata «Incentivi per favorire la diffusione dei prodotti derivanti da materiale *post*-consumo a base plastica».

chiedesse semplicemente l'estensione delle agevolazioni sul costo dell'elettricità, già in vigore per le imprese cosiddette energivore di altri settori,

acquisti in questo settore e saranno presentate con emendamenti al disegno di legge di bilancio. A questo punto, respinto l'emendamento al decreto fiscale, ci auguriamo che la convergenza che fino ad ora si

mi concentrerò su due questioni che - secondo me - hanno una grande rilevanza, contenute nel decreto fiscale al nostro esame. Premetto che voglio davvero ringraziare il relatore, Grazie di una brutta pratica, messa in campo negli ultimi anni da parte delle compagnie telefoniche e di molti gestori di servizi

Ritengo che abbiamo dato una risposta importante a 30 milioni di utenti e consumatori, e questo credo vada rivendicato. So che non è stata una partita semplice, perché le pressioni sono state molte, e ancora di più, per questo, credo vadano riconosciute al lavoro della Commissione e del relatore Lai un'attenzione e una imparzialità,

nella norma si prevedono centoventi giorni per la messa in regola, ovvero per il ritorno definitivo alla normalità: bollette ogni mese alla fine dell'anno. Da questo provvedimento - ha generato qualche discussione - sono stati esclusi i gestori delle reti energetiche, luce e gas. Evidenzio solo che, sul settore specifico, le segnalazioni di operatori che avrebbero utilizzato negli ultimi mesi il sistema dei ventotto giorni o delle quattro settimane per la bollettazione si sono molto ridotte, e comunque parliamo di servizi che si pagano a consumo, e quindi con impatto molto ridotto.

che vengano rispettati i centoventi giorni. Invitiamo gli operatori a non utilizzare tutti i centoventi giorni previsti dalla norma, perché ci si può mettere in regola molto prima e restituire correttezza al rapporto con gli abbonati. Soprattutto, chiediamo all'Agcom - è una competenza dell'*Authority* su questo versante - di procedere anche ai rimborsi di quanto pagato in maniera inappropriata - per usare un eufemismo - da parte di milioni di utenti.

nella realizzazione della metro C, di non incorrere nel rischio di perdere risorse finalizzate alla realizzazione della stessa

Per la verità, so che il Ministero di cui lei è rappresentante aveva dato parere favorevole. Si corre il rischio, però, che la bocciatura produca entro il 31 dicembre una perdita per la città di Roma di 10 milioni di euro e condizioni pesantemente anche Grazie alla relatrice sul disegno di legge di bilancio Magda Zanoni e soprattutto al Governo: varrebbe la pena di capire se ci sono spazi per recuperare quel testo.

Nel provvedimento, all'articolo 5, si prevede la parziale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l'anno 2018 mediante un minore incremento dell'aliquota, ridotta del 10 per all'11,14 per cento anziché all'11,5 com'era previsto dalla legge di stabilità del 2015. E si prevede inoltre analoga parziale sterilizzazione dell'aumento dell'accisa per l'anno 2019. Altro tema che viene rinviato per la parte corposa alla legge di bilancio è quello relativo agli enti locali e alle Regioni.

l'articolo 1‑*bis*, che prevede l'utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione per spese di progettazione. L'articolo risolve effettivamente un problema degli enti locali, perché, inserito con l'approvazione di un emendamento in sede referente, destina i proventi dei titoli abitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia anche alle spese di progettazione per le opere pubbliche. E ciò risolve davvero il problema degli enti locali, che dovevano tenere una specie di fondo a rotazione che veniva

La norma, introdotta con l'approvazione di un emendamento durante l'esame in sede referente, inserisce i fabbricati di categoria catastale A9, che sono i castelli e i palazzi di eminenti pregi artistici o storici, tra quelli che non possono essere riconosciuti quali immobili rurali agli effetti fiscali. La stessa disposizione espunge, quindi, il riferimento a quei fabbricati aventi caratteristiche di lusso.

degli enti in dissesto sarà invece oggetto di un apposito approfondimento proprio nella legge di bilancio.

E ho trovato particolarmente significativo che il Governo, fra le esigenze indifferibili, abbia fatto rientrare le modifiche alla normativa sul reato di *stalking*. l'ho trovato particolarmente significativo perché vuol dire che il Governo si rende conto dell'urgenza di

ma si dovrà andare a dibattimento. Si tratta di una contromisura attuata, perché con l'introduzione, lo scorso giugno, dell'articolo 162-*ter* del nuovo codice penale si è aperta una breccia proprio in materia di *stalking*, sembrando il reato depenalizzato tramite una condotta riparatoria, in questo caso di tipo economico. Quella che è sembrata una depenalizzazione del reato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano nel 2009, punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni, necessitava quindi di una precisazione affinché non nascessero ulteriori dubbi interpretativi.

un emendamento presentato dalla senatrice Lo Moro, assolutamente identico nel contenuto.

anche se l'imputato abbia riparato interamente mediante la restituzione in risarcimento e abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato, pur in presenza di mancata accettazione della persona offesa e anche se il giudice riconosce la congruità dell'offerta proposta. Non sarà più sufficiente procedere con un risarcimento per smacchiarsi del reato di *stalking*. Questa è certamente una misura di civiltà, che va a sanare una prassi che, se avesse continuato a perpetuarsi, non avrebbe tutelato pienamente né la dignità, né i diritti delle persone vittime del reato di *stalking*, le quali, oltre al danno, avrebbero continuato a subire anche la beffa di vedere assolto l'imputato attraverso la riparazione tramite un semplice corrispettivo economico.

un emendamento particolarmente richiesto dalle imprese locali e riguarda il diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997.

nel contesto di un provvedimento che contiene molte utili disposizioni per il Paese che puntano a metterlo nelle condizioni migliori per intercettare le positive dinamiche di ripresa, che ancora ieri ci sono state evidenziate, mi tocca l'obbligo, il dovere non piacevole ma necessario da esercitarsi, di fare una un aspetto che ritengo abbia recato al provvedimento e alle sue potenzialità un *vulnus* che temo sarà destinato a produrre effetti preoccupanti sul piano sociale e dell'occupazione, se non si troverà il modo di porvi rimedio in uno dei provvedimenti rimanenti ancora in campo in questa legislatura, a cominciare dalla prossima legge di bilancio.

per gli affidamenti che le concessionarie autostradali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono chiamate a svolgere: 60 per cento attraverso procedure di gara ad evidenza pubblica e 40 per cento per affidamenti diretti. emendamento proponeva il suddetto riequilibrio modificando la previsione attualmente vigente del codice degli appalti, che fissa quel rapporto Io vorrei sottolineare che questa richiesta di modifica, che - ci tengo a precisarlo - è stata costruita nel corso delle ultime settimane attraverso un rapporto intenso con i rappresentanti dei lavoratori e con i Ministeri competenti, e in modo particolare con i Ministeri dei lavori pubblici e dello sviluppo economico,

sull'occupazione in quel comparto, di temperare il principio con il tentativo di renderlo più graduale, attraverso un processo che poi occorrerà monitorare e rendere il più possibile incisivo. Il fatto che questo emendamento non sia riuscito ad arrivare ad approvazione ora - io lo temo e Dio non voglia che questo si verifichi - rischia di mettere immediatamente a rischio, a distanza riavvicinata, l'occupazione di

Molti di quei dipendenti e lavoratori, infatti, sono da tempo assunti con contratti a tempo indeterminato e oggi, anche nella quota che potrebbe essere recuperata attraverso il meccanismo delle gare, senza adeguati strumenti di tutela, di protezione sociale e di guida nel passaggio da un sistema all'altro, rischiano di conoscere (quelli che potrebbero essere recuperati) un percorso di precarizzazione. Come voi ben capite, per persone che hanno famiglia e un'età piuttosto significativa, ciò costituisce

un maggior rigore su un fronte che indubbiamente merita e deve essere portato a maggior trasparenza ed efficienza. Voglio però richiamare che la percentuale del 60-40 per cento è stata stabilita in uno dei

certamente Mario Monti non è uomo a cui è imputabile una particolare inclinazione a tutelare le *lobby* o a contrastare l'apertura trasparente al mercato. A questo punto rivolgo una richiesta in particolare al Governo. Governo. Avendo già provveduto a presentare lo stesso emendamento a valere sulla legge di bilancio, chiedo che tutti gli approfondimenti che probabilmente non si sono riusciti a fare in questo passaggio, e che forse avrebbero potuto fugare i dubbi residui rispetto al conflitto tra la correzione in questione e ciò che dispongono le direttive europee, vengano svolti perché il problema va portato a soluzione. sono un convinto sostenitore della necessità di portare quel sistema a trasparenza ed efficienza nel rapporto con il mercato. Ma sono anche convinto che, nel momento in cui si tratta di metterlo sulla bilancia come un passaggio probabilmente troppo rapido che il sistema non è in grado di assorbire compiutamente senza mettere a repentaglio il quadro dell'occupazione, alla fine rischia in quei termini di scaricare le sue tensioni sul fronte di quelli che sono più deboli, e cioè dei lavoratori che peraltro, costruendo nel corso degli anni un quadro di competenze professionali di notevole rilievo, vedono oggi messa in difficoltà la loro posizione. Auspico che su questo ci possano essere

credo che anche con le eventuali correzioni di quella proposta emendativa si possa trovare una soluzione, riprendendo il solco delle trattative che si sono svolte in più di un'occasione tra i rappresentanti dei lavoratori e del Governo, nelle articolazioni del Ministero delle infrastrutture che hanno fornito a quei lavoratori la rappresentazione chiara di un'apertura che oggi viene negata. E ciò ovviamente e giustamente alimenta il risentimento di quel settore lavorativo. Mi auguro che il Governo, nelle nelle successive fasi del nostro lavoro legislativo, a cominciare dalla legge di bilancio sulla quale ho presentato un emendamento, trovi lo spazio e il modo per riconsiderare il tema e portare a soluzione una vicenda che altrimenti - e e io non voglio che soprattutto noi come maggioranza di Governo ci assumiamo una tale responsabilità - rischia di produrre, per iniziativa politica del Parlamento e dell'Esecutivo, un danno all'occupazione che credo in questo momento sia l'ultimo dei prodotti che desideriamo mettere mettere sul tappeto della società italiana come lavoro di questa legislatura. *(Applausi

con il quale in tempi molti brevi si trova una soluzione a un problema che ha creato disagio a migliaia di famiglie, ai dirigenti scolastici degli istituti, al personale amministrativo soprattutto, a genitori e studenti. È un problema che nasce da una sentenza della Cassazione che ha stabilito che il coinvolgimento di un minore in un incidente fuori dal perimetro scolastico non esclude la responsabilità della scuola. Nel caso specifico, disgraziato, un bambino di undici anni era stato investito da un autobus di linea sulla strada pubblica all'uscita dalla scuola. I giudici hanno affermato e ritenuto che l'obbligo di vigilanza in capo all'amministrazione scolastica discendesse da una precisa disposizione del regolamento dell'istituto: ossia il personale scolastico aveva l'obbligo di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola le alunne e gli alunni, compresi quelli delle scuole medie. Non solo, se l'autobus fosse stato in ritardo, la vigilanza spettava al personale della scuola. La decisione, che per qualche settimana

parte del personale, che sarebbe stato sottratto da altri incarichi, con difficoltà oggettive e facilmente comprensibili. L'emendamento - come ho - come ho già detto in precedenza - risolve il problema ripristinando una regola di buonsenso, ovvero solo i genitori possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di quattordici anni dai locali scolastici al termine dell'orario di lezione. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza, e si estende, anche dopo la sollecitazione dei Comuni d'Italia, anche all'eventuale servizio del trasporto scolastico.

alla sicurezza e alla sanità. Occorre - a mio avviso - tradurre quanto contenuto nel decreto-legge per renderlo più fruibile agli uditori e ai diretti interessati, per spiegare e far comprendere in cosa si traduce nella pratica. La relazione del senatore Lai ha dato un quadro esaustivo della cornice in cui il provvedimento si inserisce: una situazione di finanza pubblica positiva con buoni livelli di crescita, con una maggiore sicurezza di poter guardare al futuro migliorando le condizioni di competitività, stimolando gli investimenti per la crescita, che si prospetta strutturale e duratura. Siamo usciti, dunque, dal *tunnel* d'inizio legislatura. Abbiamo intrapreso quella che viene definita, sempre dal relatore, un'inversione di rotta verso una decisa ripresa economica superiore alle attese. La nostra è tra le migliori crescite dei Paesi membri dell'Unione europea, con effetti immaginabili sul mercato del lavoro. Gli interventi a sostegno di piccole e medie imprese, i rifinanziamenti del fondo di garanzia, il rifinanziamento del fondo occupazione, il tema della previdenza e la regolamentazione della *cannabis* a fini terapeutici - tema ampiamente dibattuto, che ha visto un emendamento del Governo - sono alcuni dei provvedimenti più significativi. Senza entrare nei dettagli complessi dell'articolato, voglio soffermarmi, nel poco tempo concessomi - e lo ridurrò ancora, dal momento che chi mi ha preceduto ha già in parte affrontato in modo complesso il tema il tema - su alcune importanti modifiche che il provvedimento introduce per gli studenti e le famiglie. In particolare, ritengo davvero importante l'intervento sulla norma vigente che prevede, per iniziativa parlamentare, la detrazione di spesa degli affitti per gli studenti universitari che vivono oltre i 100 chilometri in un'altra Provincia. Il decreto-legge attua una modifica, con la riduzione di questa distanza, portandola a 50 chilometri per chi risiede in aree montane e disagiate, ed elimina un vincolo, quello provinciale, un vincolo davvero da superare, considerando i 100 chilometri un vincolo generale e universale, al di là della Provincia di appartenenza. È una dimostrazione davvero significativa di attenzione nei confronti degli studenti fuori sede,

emersa a seguito della recente sentenza della Corte di cassazione. Si prevede - come è già stato illustrato - la possibilità, per gli esercenti la responsabilità genitoriale, di consentire l'uscita in autonomia dei propri ragazzi dai plessi scolastici e di usufruire, sempre autonomamente, dei servizi di trasporto scolastico, esonerando, attraverso una liberatoria, il personale scolastico dalla responsabilità di sorveglianza.

e più di una tragedia, di cui sono stata anche testimone. Ricordo in particolare la tragedia accaduta all'uscita di una scuola della mia città, Gorizia, il 10 ottobre del 2000.

e drammatica per i suoi risvolti generali. Ci furono delle condanne: la maestra patteggiò otto mesi di reclusione con la sospensione condizionale e si addebitò di non aver vigilato adeguatamente sui bambini all'uscita della scuola

e zone d'ombra molto spesso i presidi scrivere circolari su circolari, per cercare di disciplinare una materia di fatto magmatica. Questo è finalmente il momento di mettere la parola fine a un drammatico problema, e le zone d'ombra saranno finalmente illuminate. un ulteriore servizio che questa legislatura ha reso alla scuola e alla famiglia, per una buona interrelazione tra le componenti fondamentali del nostro sociale.

Intendo intervenire su un articolo che si propone di inserire nel testo originario, precisamente sull'articolo 19-*bis*, che riguarda l'equo compenso e le clausole vessatorie. Nell'ambito di tale articolo sono stati inseriti due punti estremamente importanti e rilevanti per il mondo sanitario e per l'impatto positivo che avranno sulla pubblica amministrazione. Il primo punto prevede che le disposizioni di cui all'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si applichino, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e, quindi, ai professionisti sanitari, anche iscritti a ordini e collegi, i cui parametri sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27. Questa apertura, come accennavo, è considerata molto importante - e lo è davvero - perché rende dignitoso il lavoro di tanti professionisti sanitari che operano in qualità di liberi professionisti nei rapporti convenzionali aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cura, di assistenza e di riabilitazione. definizione che è stata inserita nell'articolo 19-*bis*, che è considerato tale quando risulta proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione sanitaria, assistenziale e riabilitativa, è assai

un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista sanitario. che consentono di poter utilizzare le norme inerenti all'equo compenso anche in ambito sanitario e che riguardano un numero significativo di professionisti. Faccio solo un esempio, senza voler allargare la considerazione, agli oltre 30.000-35.000 infermieri liberi professionisti che apprezzano molto questa definizione; ma soprattutto, oltre ai liberi professionisti, penso ai fruitori delle prestazioni di questi professionisti (infermieri, tecnici della riabilitazione, tecnici sanitari di diversa qualifica e funzione, che erogano le loro prestazioni sanitarie assistenziali direttamente ai cittadini), che potranno contare su un'impostazione assistenziale strutturata con efficacia e appropriatezza ed entro un *range* temporale

rendendola inefficace, inappropriata e tesa solo all'utilizzo del minor tempo possibile per cercare di stare dentro un compenso che equo non è. È infatti noto come, per garantire i servizi di cura e di assistenza, fermi restando i vincoli assunzionali, molte aziende e strutture sanitarie, soprattutto quelle private, si avvalgano di professionisti regolati da rapporti convenzionali per l'effettuazione di prestazioni estremamente delicate, delicate, che si vedono, quindi, mal definiti e mal compensati rispetto alle prestazioni che eseguono. Teniamo conto che buona parte delle strutture sanitarie, soprattutto del privato e del privato convenzionato, utilizzano queste forme di

che hanno depauperato in maniera significativa le strutture del servizio sanitario pubblico, oltre che quelle sanitarie private; ma non solo: anche le strutture sociosanitarie

la struttura portante, il nerbo, del nostro servizio sanitario e socio-assistenziale, che si rivolge direttamente ai cittadini. Credo quindi che attraverso l'inserimento dell'articolo 19-*bis* e, soprattutto, di questa apertura, che non riguarda più solo gli avvocati, ma anche tutti gli altri

la partita fiscale con l'insieme dei provvedimenti e della struttura degli interventi nel nostro Paese, devo dire con soddisfazione, anche nel campo del *welfare*. Ciò non era scontato.

non necessariamente di carattere monetario diretto, ma anche attraverso la leva fiscale.

Il fatto di avere un contesto favorevole anche per quel che riguarda il *deficit* pubblico sotto controllo ci consente e ci ha consentito di aprire ad alcune questioni che sono state da noi evocate

Voglio iniziare esprimendo soddisfazione per l'emendamento che riconosce la detraibilità degli alimenti a fini speciali;

di patologie e di malattie rispetto alle quali è sempre molto difficile intervenire, se non in termini strettamente assistenziali. In questo caso noi riconosciamo

Provate una volta a non riuscire a ingoiare; è una cosa terribile e lo è in particolare nelle fasi terminali dell'esistenza. Tutta questa parte è ricompresa nella defiscalizzazione. Concordo con il Governo che in via sperimentale perché c'è un problema di comprendere anche la platea e gli effetti. Non ci sono assolutamente problemi, ma voglio dire che oltre al segnale strettamente economico e fiscale, vedo un segnale etico

abbiamo una combinazione virtuosa, che consente interventi che, mi auguro, possano essere realizzati su tutto il territorio nazionale in modo omogeneo, accanto ad interventi individuali e quindi alla possibilità della singola persona, del del singolo malato e del singolo paziente di poter agire sulla leva fiscale per affermare un suo diritto. Questo è poco? È tanto? Io trovo che sia straordinario e credo che ne dobbiamo andare tutti davvero molto fieri. Se leghiamo questo elemento all'altro importante lavoro sulle neuroscienze (non solo l'adroterapia, ma - in generale

si fa sempre fatica a intervenire. In questo caso, abbiamo aperto con il Governo una pista molto importante e spero che potremo andare avanti in questa direzione anche per quanto riguarda un incremento ulteriore della ricerca

dei problemi rilevanti, di cui abbiamo discusso in quest'Aula. Il primo problema rilevante è che si tratta di un farmaco e, quindi, come tale deve essere sottoposto a tutti i percorsi di sicurezza che il farmaco richiede. È per questo che il lavoro fatto dall'altro ramo del Parlamento ha consentito di mettere a sistema un intervento che

vorremmo pensare che debbano andare a procacciarsela da qualche parte in modo illegale. Quindi, è giusto e sacrosanto che, nella massima sicurezza, si possa procedere In secondo luogo, è importante che come Parlamento abbiamo integrato l'emendamento del Governo, aggiungendo un'altra possibilità

l'infiorescenza della *cannabis* che potremmo produrre tranquillamente essendo il nostro, come noto, un Paese che ha nulla da invidiare all'Olanda, tantomeno al Canada per quanto riguarda il sole. Quindi, il punto non è se si coltiva o no, ma se ci sono le garanzie della sicurezza

Colgo l'occasione anche per augurarmi che molto presto possa andare in votazione la delega al Governo, in terza lettura al Senato, che riconosce le professioni sanitarie, di cui abbiamo bisogno per impedire l'abusivismo sanitario e per riconoscere la dignità professionale a queste persone, anche nel campo della sanità. L'equo compenso è anche questo: evitare che

nel passaggio tra pubblico a privato e nelle diverse situazioni di questo Paese. L'equo compenso rimane uno dei punti di riferimento. Il secondo elemento che vorrei citare riguarda l'emendamento che abbiamo presentato sulla Croce Rossa. di un dibattito importante e voglio semplicemente segnalare che la nostra posizione non è pregiudizialmente contraria a nulla, ma abbiamo voluto segnalare dei problemi, che obiettivamente esistono, in una fase di transizione del modello

per quel che riguarda gli assetti patrimoniali, il futuro del personale e il tipo di intervento che un organismo così importante svolge nel mondo. Il Governo ha avuto un'altra posizione e ne prendo atto molto tranquillamente. L'ultima questione, che riguarda

disegno di legge di riordino delle attività funerarie nel nostro Paese. C'è un problema molto grande di correttezza e di trasparenza su attività fondamentali, che sono ormai imprenditoriali, anche di un certo livello, che richiedono trasparenza chiarezza di regole e anche che i cittadini possano non sentirsi oberati in un momento così tragico, come la scomparsa di una persona cara.

nella legge di bilancio si possa individuare almeno uno spazio che ci consenta di arrivare ad una riforma dell'intero sistema, di di cui c'è molto bisogno dal punto di vista sanitario e imprenditoriale e dal punto di vista della correttezza dei rapporti con i cittadini. Voglio terminare il mio intervento con un augurio al Governo, che sostengo e quindi anche ciò che mi piace un po' meno lo accetto lo stesso, perché ritengo sia molto importante che il Governo possa andare avanti e terminare un lavoro davvero straordinario.

chiarire a questa Assemblea di cosa si tratta. Finalmente il Governo ha definito lo stato giuridico degli *ex* emigrati, ed *ex* frontalieri, cittadini che hanno lavorato per un periodo all'estero, iscritti all'AIRE, che sono rientrati in Italia, e sono diventati, per colpa di un "danno collaterale" nella denuncia volontaria dei capitali detenuti all'estero, degli evasori.

Tutto a un tratto, con la dichiarazione volontaria, sono diventati evasori. A dire il vero, noi senatori del collegio estero questo problema lo avevamo segnalato nella fase di discussione della

persone, a dimostrazione che nello stesso Governo la capacità di ascolto di un componente o di un altro può portare a una soluzione o non soluzione.

«sanatoria» o «condono», anche se tecnicamente somigliano a questo, non c'entrano assolutamente nulla. Devo però anche cogliere l'occasione per lasciare agli atti di questa Assemblea che un problema resta, Vice Ministro. L'emendamento risolve totalmente il problema di chi già è rientrato in Italia o rientrerà da qui al 31 luglio 2018.

però - fatemelo dire un po' scherzosamente - considerando che mi auguro di finire la mia vita in Abruzzo, se rientrerò nel 2019, già oggi so che rientrerò da evasore fiscale. Questo va chiarito con una norma strutturale dopo questo passaggio; vorrei semplicemente che questo aspetto restasse agli atti, e che nella prossima legislatura, se non sarà possibile farlo adesso, venisse chiarito definitivamente.

Abbiamo ridotto notevolmente i finanziamenti ai patronati in questi anni creando loro problemi di liquidità. Abbiamo quindi fatto una proposta, Vice Ministro, per aumentare l'acconto. Posso capire che questo porta a un bisogno di cassa supplementare, però il bilancio complessivo dello Stato non aumenta di un euro. Dunque, uno sforzo per dare loro un acconto superiore, per poterli almeno sgravare dai dai costi bancari, credo sia necessario. Ho fatto un rapporto che solleva problemi nel funzionamento dei patronati all'estero, ma sono istituzioni importanti per le nostre comunità. Mi auguro che il Ministero del lavoro legga il rapporto che il Comitato

Dunque i patronati vanno riformati e rivisti, ma vanno soprattutto messi in condizioni di operare. Faccio qui un appello affinché nella legge di stabilità si possa dare una risposta positiva alla legittima richiesta che proviene dai patronati. L'ultimo punto molto specifico,

una norma fiscale retroattiva che abbiamo introdotto con il decreto salva Italia tre anni fa: una norma assolutamente scorretta, per la quale i tribunali italiani ci stanno condannando, ci stanno condannando, che non siamo mai riusciti a correggere e ha già portato alla morte di piccole imprese, fatte da italiani all'estero, che avevano come principale responsabilità quella di promuovere il turismo verso

e credo che sia un dovere minimo da parte nostra quello di correggere la norma. Caro Vice Ministro, l'ho ringraziata prima e la ringrazio ancora, perché so che di questa storia lei

di sospensione - dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso, appunto, tra il 9 settembre e il 30 settembre 2017. sospensione e non ovviamente di esenzione, vale a dire che le mancate entrate erariali per il 2017 vengono recuperate nell'anno successivo. In termini tecnici è un differimento della riscossione. Nella tabella allegata al provvedimento di analisi degli impatti si riporta correttamente che i 55 milioni ipotizzati dall'impatto della misura, stimati

alla sola città di Livorno e ai soli residenti che erano in possesso di dichiarazione di inagibilità della propria abitazione, inagibilità riconosciuta dall'autorità competente. Il provvedimento così formulato limitava l'intervento Paradossalmente - questo è l'aspetto su cui si è determinato il disguido - per i comuni limitrofi di Collesalvetti e Rosignano, Rosignano, toccati più marginalmente dall'evento, la stessa misura era estesa indistintamente a tutti i residenti. Con ogni evidenza la misura risultava ingiustamente squilibrata,

ha esteso il criterio, originariamente previsto per il comune di Livorno, anche ai confini di Collesalvetti e Rosignano, di fatto vanificando l'intera misura, restringendola cioè alle sole 35 persone di Livorno. Vorrei, Vice Ministro, relatore, che fosse chiaro: i danni nella città, nel Comune di Livorno sono stati davvero ingenti e diffusi, anche se non necessariamente

fosse concessa a coloro che avessero subito gravi danni riscontrati e appurati dall'elenco predisposto dal Commissario per l'emergenza e sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della protezione civile. Era sostanzialmente una misura di riequilibrio

Chiaramente, anche per il ruolo che immeritatamente rivesto, direi che nei minuti che mi rimangono voglio però intervenire anche sulle misure e sugli interventi previsti da questo collegato attinenti alle politiche dei trasporti e devo dire, signor Vice Ministro, manifestando davvero un sincero e convinto apprezzamento, a partire dall'articolo 12, di cui non mi è sembrato che nella discussione generale vi sia stata in qualche modo alcuna segnalazione. Mi riferisco ovviamente al provvedimento inerente all'Alitalia, provvedimento a mio avviso di grande intelligenza e lungimiranza politica, per svariati motivi che brevemente voglio tratteggiare. In primo luogo, perché stabilizza l'attuale, delicatissima situazione che rispetto al passato - vorrei sottolineare - è sicuramente meno grave e più interessante, con novità cui appunto voglio accennare. In primo luogo, finalmente si assiste ad un *management* competente e serio. dottor Gubitosi, contrariamente a quello che è avvenuto nel passato anche recente (mi riferisco alle numerose esperienze che si sono susseguite, dai "capitani coraggiosi", ai francesi, agli arabi) mi sembra che oggettivamente si stia facendo sul serio, cioè si interviene sulla struttura di Alitalia, modificando i contratti in essere e determinando risparmi che da tempo segnalavamo assolutamente opportuni.

eliminare quell'elemento di imbarazzo e di precarietà che ne poteva derivare. Vi è da aggiungere, per capire anche la situazione delicata ed interessante - non delicata e grave - che abbiamo registrato, negli ultimi mesi, insieme all'opinione pubblica, anche le difficoltà che stanno attraversando le compagnie *low cost* e credo che questo aspetto possa consentire di guardare in modo nuovo, superando un certo strabismo che le politiche di governo a tutti i livelli hanno avuto per le compagnie *low cost*, perché in molti casi hanno determinato fortuna e sviluppo di scali minori

Questi due aspetti - un *management* competente e serio, che ha messo per la prima volta le mani in maniera adeguata sulla struttura di Alitalia, negoziando anche contratti capestro e producendo risparmi, in combinato disposto con le difficoltà delle compagnie *low cost* - hanno determinato non a caso anche nuove offerte sia da soggetti americani sia il rinnovo delle offerte da parte delle compagnie tedesche.

sulla prossima - ma già in corso - campagna elettorale. Credo che questo intervento abbia sicuramente contribuito ad evitare il ripetersi della campagna

e non fare presto; perché in questa fase fare presto o fare tanto per fare può implicare soltanto fare male. Voglio infine felicitarmi davvero con la Commissione e con il Governo anche per il lavoro che è stato fatto nelle ore notturne su altri provvedimenti, con gli ulteriori emendamenti approvati. Come leggevo nel Resoconto, sul trasporto aereo

sugli aeroporti e sulle infrastrutture aeroportuali si prevede sostanzialmente che il concessionario in scadenza di concessione e in grado di intervenire con gli investimenti necessari non debba essere costretto a non intervenire perché magari non gli possono essere riconosciuti. Sono provvedimenti minimi che passano sotto silenzio, ma che a mio avviso hanno davvero la funzione di liberare risorse private per investimenti di utilità pubblica.

in Puglia. Ebbene, questo provvedimento, molto articolato, molto importante e molto serio, non stanzia solo risorse ma prevede l'intensificazione dei controlli, l'assunzione di personale per quanto riguarda l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, interviene su una temporalizzazione che rende credibile le risorse assegnate e prevede parimenti anche controlli di verifica

Vice Ministro, onorevoli senatori, prima di svolgere valutazioni generali desidero entrare subito su un tema preciso che al sottoscritto e al Gruppo parlamentare di Forza Italia sta molto a cuore. I dati non lasciano spazio ad interpretazioni. I liberi professionisti e i lavoratori autonomi in Italia sono 1,3 milioni e rappresentano per numero e per ricchezza prodotta sicuramente una categoria indispensabile per la crescita dell'intero Paese. Purtroppo però in Italia l'iniziativa autonoma nel campo del lavoro non viene adeguatamente sostenuta, ma al contrario spesso viene ostacolata dallo Stato. Questi ostacoli ahimè - vanno rimossi al più presto, a partire dall'eccessiva pressione fiscale e dall'asfissiante ragnatela burocratica che attanaglia purtroppo le aziende. Inoltre, in riferimento al provvedimento al nostro esame, ci siamo battuti con emendamenti specifici per introdurre l'equo compenso, perché è nello stesso interesse dei cittadini essere supportati da professionisti competenti e qualificati, mentre la corsa al ribasso del costo delle prestazioni fa sicuramente scendere anche la qualità dei servizi offerti e, di conseguenza, la soddisfazione dei cittadini. Questo tema è stato inizialmente stralciato dalla manovra, ma abbiamo insistito che si affrontasse perché riveste una importanza tale da non poter essere sottaciuto. Prendiamo atto con soddisfazione che il Governo ha riconosciuto in Commissione bilancio la validità delle nostre argomentazioni, inserendo un emendamento per l'introduzione dell'equo compenso, è purtroppo solo parziale perché, se ci si fosse mossi in tempo, avremmo potuto fin da ora migliorare il testo affinché potesse soddisfare a pieno le legittime aspettative di tutti gli ordini professionali e non. Ritornando su un piano più generale, la manovra di bilancio approdata al Senato contiene diversi elementi che meritano quanto meno un'analisi approfondita. Il primo ha senz'altro a che fare con i numeri, cioè con la dimensione complessiva degli interventi previsti: abbiamo visto che su un totale di circa 21 miliardi di euro, ben 14,9 sono destinati ancora una volta a evitare l'applicazione degli aumenti dell'IVA imposti dall'Europa a garanzia della tenuta dei conti pubblici. Com'è ben noto, a causa degli impegni presi dal nostro Paese in sede europea, sono state da tempo introdotte le cosiddette clausole di salvaguardia a garanzia del rispetto del percorso di rientro dei nostri conti pubblici. Le clausole più pesanti riguardano proprio l'aumento automatico dell'IVA per permettere allo Stato di avere maggiori introiti e possono essere neutralizzate solo con altre opportune misure. Anche quest'anno, infatti, quasi 15 miliardi di euro di maggiori entrate e di minori spese sono finalizzati soltanto a rispettare un obbligo contabile, frutto degli accordi europei, di cui ormai però sfuggono le motivazioni, come osservato da diversi economisti. Oggi siamo qui a discutere di una manovra che nel suo complesso rischia seriamente di compromettere i timidi segnali di ripresa in atto della nostra economia. Parlo di timidi segnali, non per mancanza di ottimismo. Se non fossi ottimista non potrei fare l'imprenditore, perché fare impresa in Italia è quasi un gesto eroico, vista la tassazione e la burocrazia che bisogna sopportare. Sono i numeri che parlano chiaro: 1'Italia ha sprecato la ripresa economica che ha interessato tutta l'Europa. Secondo il Fondo monetario internazionale (FMI) il PIL in Europa aumenterà del 2,4 per cento nel 2017, mentre in Italia appena dell'1,5 per cento. Nel prossimo anno andrà pure peggio, perché si prevede un aumento del PIL italiano di 1,1 per cento, mentre quello europeo sarà +2,1 per cento. Siamo e restiamo sempre più fanalino di coda in Europa. La nostra economia è la più debole, segno inequivocabile della politica inefficace dei Governi di centrosinistra di questi anni. Domandiamoci quindi: l'odierno stato di salute dell'economia della zona euro e quello dei nostri conti giustificano una manovra come quella presentata oggi dal Governo? Onorevoli colleghi, ad esaminarla, questa manovra, pare in gran parte niente altro che una pesante partita di giro, in cui si scongiura un aumento dell'IVA imposto dall'Europa praticando tagli tagli reali, tuttavia essa rischia di non soddisfare il giudizio della stessa Unione europea, come ieri ha detto il Vice Presidente della Commissione europea: è evidente, infatti, che 15 miliardi su 21 non produrranno sicuramente effetti positivi. Vorrei ora brevemente soffermarmi su ciò che resta, tolti i già citati 15 miliardi di euro, e ancora una volta mi pongo e vi pongo un interrogativo: quali scelte in ambito di politica economica si possono fare, dal momento che la parte vera della manovra ammonta a meno di 6 miliardi? Mi sembra fin troppo ovvio che, alla luce di questi numeri, operare scelte significative, in grado di ridare slancio al sistema Paese, risulta impresa pressoché impossibile, tanto più che quasi la metà della cifra effettivamente stanziata (circa 3 miliardi di euro) è finalizzata al rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici. Scorrendo i 120 articoli che compongono il testo della manovra, non ho trovato una sola riflessione significativa sui temi fiscali, mentre nel decreto fiscale ad essa collegato l'unico dato rilevante è l'ennesimo rinvio di un miliardo di aumenti dell'IVA, recuperando ulteriori entrate. Ma appunto solo di un rinvio si tratta, che significa lasciare - ahimé - questa spada di Damocle In compenso si perpetua la politica dei *bonus* a pioggia, con criteri che alcune volte sfuggono a qualsiasi logica. Abbiamo allora l'allargamento della platea dei beneficiari degli 80 euro, l'inserimento del *bonus* per gli abbonamenti autobus, treni regionali e metro, la proroga del *bonus* cultura per i diciottenni, dell'ecobonus per le ristrutturazioni edilizie, del *bonus* giardini, dello sconto del 19 per cento sulle polizze anticalamità sulla prima casa e altri *bonus* ancora. Da un lato, dunque, si rimanda la soluzione di problemi essenziali, preferendo lasciarla ai posteri, come l'aumento dell'IVA; dall'altra si insiste con misure *una tantum*, pescando soldi dalla fiscalità generale. Tralasciando per un momento la dubbia efficacia di simili interventi, ci pone di fronte anche ad una evidente contraddizione, perché la fiscalità generale dovrebbe privilegiare interventi di matrice strutturale e soprattutto volti a rispettare il principio costituzionale della progressività, per cui i benefici di natura pubblica dovrebbero essere destinati essere destinati alle fasce socialmente più deboli e non spalmati in maniera uniforme sull'intera platea della popolazione. Ovviamente, a nessuno qui sfugge la ragione di tali scelte: è senz'altro più semplice distribuire soldi a pioggia, che elaborare politiche di sostegno socioe-conomico più mirate e senz'altro garantisce maggiore visibilità politica, soprattutto con l'avvicinarsi della campagna elettorale. Tuttavia, le istituzioni non sono chiamate a fare Anche quando sono state introdotte misure giuste, come il rifinanziamento del credito di imposta per le imprese, le risorse ci sono apparse insufficienti, specie al Sud, se pensiamo che i fondi stanziati per l'industria 4.0 sono solo il 10 per cento dei 14 miliardi stanziati alle imprese di tutta la Nazione. Al Governo chiedo: che ne è delle promesse di taglio del cuneo fiscale e degli altri interventi annunciati per rendere più pesanti le buste paga dei lavoratori e meno onerose le assunzioni stabili? Anche per queste ragioni, e concludo, la manovra 2018 e il decreto fiscale ad essa collegato pongono un'ipoteca sul futuro di questo Paese, di cui la maggioranza di questo Parlamento si assume tutta la responsabilità.

Signor Presidente, intervengo in sede di discussione generale sul decreto-legge collegato alla legge di bilancio innanzitutto per segnalare un fatto che appare di evidenza solare: questo decreto-legge, che negli annunci e nei proclami di Governo avrebbe dovuto interessare *in primis* l'annosa questione della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia, ovvero il reperimento di risorse per evitare l'innalzamento delle aliquote IVA, ne contiene solo un timido accenno poiché, di fatto, la questione viene rinviata alla legge di bilancio. misura è chiaramente condivisa, ma la domanda sorge spontanea: allora perché questo decreto-legge è stato emanato? Nelle norme sottoposte al nostro esame non si ravvedono evidenze di necessità e urgenza e l'omogeneità, requisito di ogni decreto-legge, è palesemente inesistente. La semplice verità è che vi siete assunti la responsabilità di emanare un decreto-legge che contiene solo le vostre urgenze e quelle delle parti politiche che vi sostengono. Mi riferisco, ad esempio, alla norma che stabilisce la proroga per la cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia, dal 30 aprile 2018 al 30 settembre 2018. La filosofia di fondo è: problema rinviato, mezzo risolto. si spendono altri denari pubblici, ben 300 milioni di euro, decisamente troppi, ma tanto paga Pantalone. E Pantalone è rappresentato da tutti quei cittadini vessati che tirano la carretta per tutti e non ne possono più. Il tutto avviene per consentire una sorta di corteggio affaroso tra chi sostiene di voler acquistare e chi deve vendere. È doveroso garantire la continuità del servizio di trasporto aereo fino all'effettivo trasferimento dei complessi aziendali, ma, di posticipo in posticipo, Alitalia non verrà mai ceduta in tempi non dico celeri, ma nemmeno ragionevoli, sottraendo risorse importanti per altri servizi pubblici parimenti necessari. In alternativa, si renderà necessaria un'ulteriore imposizione fiscale. In entrambi i casi, i cittadini sapranno come ringraziarvi: con il voto. Chi è causa del suo mal, pianga se stesso. Questo Paese non può permettersi altre tasse. La Corte dei conti, centri di studi economici internazionali e tutte le persone di buonsenso sottolineano come il nostro Paese sconti un eccessivo carico tributario. L'OCSE classifica l'Italia al quinto posto tra i Paesi europei per imposizione fiscale per singolo contribuente e siamo sul podio, al terzo posto, per le famiglie monoreddito. Questa condizione non consente di certo alle famiglie, soprattutto a quelle più esposte alla crisi economica, quelle più bisognose, di nutrire rosee speranze nel futuro e senza le famiglie non avremo un futuro. Avete trasformato le agenzie fiscali in enti bramosi di lucro che lavorano a provvigione (0,823 per cento dell'incasso per l'Agenzia delle entrate e 1,338 cento dell'incasso per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli), mentre stiamo parlando di pubblica amministrazione e non di un'azienda privata. Dove è la terzietà a garanzia del cittadino contribuente? Una pubblica amministrazione deve coprire le spese e non generare utili. L'Italia è un Paese dove certe aziende private scaricano il loro rischio di impresa sui cittadini e dove la pubblica amministrazione fa profitti facendo cassa sul cittadino come fosse un'azienda privata. siamo riusciti ad applicare, in barba ad ogni principio costituzionale, le imposte sulle tasse, vedi l'IVA applicata alla TIA, quindi l'IVA applicata ai tributi, oltre che alle tariffe. Possiamo ben comprendere che il cittadino non è visto come un utente cui rendere un utile e e dignitoso servizio, ma come un limone da spremere. E, proprio come un limone spremuto non può più dare succo: un cittadino vessato porta poi anche lo Stato necessariamente a un periodo di secca. Mi diranno che semplifico: certamente. Diciamo che per me questo è l'unico modo per cercare di capire concretamente ciò che appare fumoso, contorto, privo di senso e, a ben guardare, lesivo per tutti. Probabilmente, l'unica vera urgenza del Governo è stata quella di esercitare il cosiddetto *golden power* su Telecom Italia. Purtroppo il bel Paese è divenuto terra di conquista per investitori stranieri. Le nostre migliori imprese, quelle che ci hanno resi grandi e noti nel mondo (anche grazie al *brand made in Italy*, che è il terzo per importanza nel mondo), troppe volte non sono più nostra proprietà. Tralascio considerazioni di ordine più generale sulla necessità di regolamentare i tempi della globalizzazione selvaggia e la libertà di impresa, per concentrarmi su imprese strategiche. Di certo la presenza incombente di Vivendi, ormai azionista di maggioranza di Telecom, è stata determinante per l'emanazione di questo decreto-legge. Più che estendere il *golden power*, il Ministro competente avrebbe dovuto mettere il Paese al riparo dai rischi, scorporando Sparkle, il ramo d'azienda che detiene la rete infrastrutturale (per intenderci, quella che detiene la proprietà dei cavi sottomarini che garantiscono le nostre comunicazioni e che collegano l'Italia al resto del mondo), e Telti, la società che fornisce servizi *software* grazie ai quali vengono prodotte le comunicazioni sensibili anche tra enti governativi. Questo decreto-legge, più che motivato dall'urgenza, è pregno di fretta per il tanto tempo perso, visto che il necessario da farsi era noto da tempo. Nella società 4.0, dell'industria 4.0 e della cultura 4.0, non possiamo perdere il controllo delle reti. La proprietà delle reti deve deve rimanere monopolio naturale dello Stato e garanzia di fondamentali interessi comuni. Una misura giusta, doverosa e attesa, già discussa in Commissione lavoro e da me depositata l'8 marzo, ma - perdonate l'immodestia - ben più organica, strutturata, compiuta, sottoscritta da tutto il Gruppo Federazione della Libertà, l'equo compenso riafferma la dignità dei liberi professionisti. Si tratta di una questione di rispetto delle competenze e delle professionalità, un doveroso allineamento della legge con i principi di uguaglianza e universalità tra tutte le categorie professionali. Lavoratori da tutelare soprattutto nel caso di commissioni da rendere ai cosiddetti contraenti forti, a iniziare dalle pubbliche amministrazioni. Una misura che argina la guerra al ribasso delle parcelle professionali, tutela la qualità della prestazione del servizio reso, nonché la trasparenza e la congruità del costo per il cliente committente. Si era detto tante volte, ma vi siete mossi solo dopo le manifestazioni di piazza. Avete tirato fuori il populismo che è in voi. Ebbene, una norma così importante avrebbe meritato altro tempo, una maggiore decantazione e una maturazione, come ammesso dallo stesso collega Lai. Una norma importante fatta alla carlona,

avente per di più, in prospettiva elettorale, lo spirito del milleproroghe. Dentro ci avete messo di tutto, pure le norme che consentono di lasciare i ragazzi liberi di tornare a casa da soli, norme che non sarebbero mai neanche dovute essere ipotizzate.

sulla tanto attesa liberalizzazione del mercato della gestione dei diritti d'autore, attraverso la piena attuazione della direttiva 2014/26/UE. Su questo tema il Governo ha reiterato una serie infinita di no, nonostante i numerosi atti di sindacato ispettivo, emendamenti proposti trasversalmente e gli ordini del giorno approvati. Un no, si diceva, «consentito dalla normativa UE, che è pienamente legittimo». Una direttiva, che doveva essere recepita entro il 2016. Abbiamo bucato questo termine perché, secondo il ministro Franceschini, era necessario riflettere di più sul corretto recepimento. E così, tentennando, perché non si ha il coraggio di affrontare seriamente i problemi e risolverli, il 30 maggio 2016 ci è stato notificato l'avvio di una procedura di infrazione. Il pomo della discordia è l'articolo 5 della direttiva Barnier, il diritto di scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva al quale affidare la gestione delle proprie opere. Perfino l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il 10 giugno 2016, ha formulato una serie di osservazioni volte ad un recepimento più coerente della direttiva, sollecitando l'intervento di liberalizzazione integrato da una riforma complessiva delle modalità di intermediazione dei diritti delineate dalla legge sul diritto d'autore, rivedendo il ruolo e la funzione della SIAE. Nulla di fatto. Si è deciso di mantenere in vita l'articolo 180 della legge sul diritto d'autore, lasciando intatto il monopolio della SIAE. La risposta a tutte queste richieste è stata, più o meno indirettamente: il monopolio non si tocca perché l'Europa non lo chiede. Peccato che poi il ministro Franceschini e il sottosegretario Gozi, nella splendida cornice del festival del cinema di Venezia, si siano sentiti chiedere dal commissario europeo per l'economia e la società digitali Gabriel

pianga se stesso. I carrozzoni vi piacciono troppo, fanno parte del vostro DNA. Le complicazioni sono la normalità del vostro procedere, come è accaduto nel sisma, dove le cose buone finiscono senza esito positivo: 6 decreti-legge con la stabilità, 41 ordinanze ed ora servono le linee guida. Risultato? Il nulla. Un *to be tra Ceriscioli e la commissaria per il terremoto De Micheli, che non porterà a nulla. Nelle Marche abbiamo un Presidente che si limita a sorridere inutilmente. anticipato 700 milioni del miliardo di euro dell'Unione europea: inservibili, come dare il pane e togliere i denti. Sempre perché siete l'ufficio complicazione cose semplici, avete bocciato un emendamento che proponeva una sanatoria degli avvisi bonari all'Agenzia delle entrate. Semplice buon senso, in armonia con la rottamazione delle cartelle, ennesima prova del nove su quanto poco buon senso e nessuna logica regni in queste consunte Aule. Abituati ad usare un neurone isolato per volta, come la particella di sodio nell'acqua Lete, come Orlando che aveva applicato l'equo compenso ai soli avvocati senza condividerlo alle altre professioni. Eppure le sinapsi sono le autostrade della conoscenza, dell'esperienza e della saggezza che dimostrate di non avere. Un Paese che vuole crescere deve guardare i Paesi che stanno già crescendo, come la Spagna e l'Irlanda, dove ci sono futuro e occupazione grazie all'affidabilità del bilancio. futuro, debiti limitati e riforme. Questa frase non è mia, è di Manfred Weber, colui che ha detto a Renzi di non frignare e si è augurato la vittoria elettorale di Berlusconi. "Il link apre una nuova finestra") *(LN-Aut)*. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio consente di fare un resoconto di fine legislatura delle politiche di questa maggioranza, sempre più dilaniata da scontri interni. Il relatore Lai, che ringrazio per la disponibilità nel lungo e intenso lavoro fatto in Commissione, nella relazione di stamane ha ovviamente, da senatore del PD, decantato la *policy*, le politiche economiche messe in campo dal Governo Renziloni e dai due che l'hanno preceduto (Letta e poi Renzi). Ha parlato di inversione di rotta, di maggiore competitività del Paese, di equilibrio economico nei conti pubblici. Ebbene, vorrei ricordare che le cose non stanno proprio così. Lo sanno gli oltre 7,5 milioni di italiani in stato di deprivazione, di cui 4,5 milioni in povertà assoluta; lo sanno gli italiani - sempre più numerosi - che rinunciano alle cure perché non hanno soldi per le medicine e per fare gli esami; lo sanno i tanti disoccupati, soprattutto i tanti giovani, che non trovano lavoro, anche perché sempre più attività economiche chiudono per la crisi e, talvolta, anche per l'eccesso di credito nei confronti della pubblica amministrazione, che non paga. A proposito, aspettiamo ancora che Renzi salga a piedi sul Monte Senario, visto che ha bucato clamorosamente l'ennesima promessa. Lo sanno i tanti, tantissimi italiani, oltre 120.000 l'anno, in gran parte giovani diplomati e laureati, che, non vedendo prospettive, preferiscono emigrare all'estero, magari a fare i camerieri a Londra o a Parigi. No, le cose non vanno affatto bene! E questo nonostante il contesto europeo e mondiale favorevole: il *quantitative easing* di Draghi, gli interessi bassi del costo del denaro e il basso costo del petrolio. Noi cresciamo, ma poco e in misura molto minore rispetto agli altri Paesi d'Europa. Peggio di noi sta solo la Grecia. Anche i dati odierni dell'ISTAT lo dimostrano: la produttività del lavoro è scesa dell'1 per cento nel corso del 2016, dopo gli aumenti degli anni precedenti. Anche il divario tra la nostra disoccupazione e la media dell'Unione europea sta aumentando. E che dire del nostro debito pubblico? A settembre ha registrato quota 2.283,7 miliardi, più 177 miliardi rispetto a febbraio del 2014, mese in cui si è insediato Renzi a capo del Governo. D'altronde, che siamo in difficoltà lo certificano i numeri magri della legge di bilancio: tre quarti della manovra di poco più di 20 miliardi sarà impiegata per neutralizzare le clausole di salvaguardia introdotte dal Governo Letta, cioè evitare un catastrofico aumento dell'IVA. Ci sono pochissimi investimenti, non solo per nuove infrastrutture, ma anche per le manutenzioni. Ci sono poche misure per la crescita, per il contrasto alla povertà e per il sostegno alle famiglie. E che dire delle coperture? I risparmi derivanti dalla *spending review* che si tradurranno in altri tagli lineari a Regioni, e soprattutto, ai Comuni; 5 miliardi sono previsti dalla lotta all'evasione fiscale, ma qui vi è però un'enorme incertezza assoluta, come hanno sottolineato giustamente la Corte dei conti e l'Ufficio parlamentare di bilancio; e poi, per concludere la copertura, oltre 10 miliardi sono nuovo debito pubblico: tanto, su 2.300 o quasi, questi incidono poco. Nel merito del decreto-legge tocco due o tre aspetti. Sulle calamità naturali, il provvedimento solo dopo l'esame affronta, ma non tutti, i problemi aperti legati soprattutto al *post* emergenza e ricostruzione del terremoto del Centro Italia dello scorso anno. Si occupa però, o tenta di occuparsi, anche dei sismi dell'Emilia-Romagna e della Lombardia del 2012, dell'Aquila del 2009, dell'Umbria del 1997 e di quello recente di Ischia. All'emanazione, però, lo ricordo, il decreto-legge si occupava solo poco più che dell'alluvione di Livorno. Poi, viste le centinaia di emendamenti trasversali che portavano le tantissime e disperate istanze dei terremotati, soprattutto dal Centro Italia, si è deciso di metterci seriamente mano.

e sono SAE che registrano dei costi esorbitanti. In termini di macerie, ne sono state rimosse solo il 10 per cento. E così è arrivato

Purtroppo, pur riconoscendo la buona volontà del neo commissario alla ricostruzione De Micheli, tanti problemi restano aperti e non vengono date risposte a tante esigenze. Come, per esempio, quelle del Comune di l'Aquila, la cui nuova amministrazione, che si è insediata nella scorsa primavera, ha trovato da quelle parti un disastro totale e molta polvere sotto il tappeto. Certo, siamo anche riusciti a ottenere cose positive. Per esempio su nonna Peppina, simbolo degli sfollati, è bene che il Governo abbia recepito la richiesta della Lega che, dopo aver depositato un disegno di legge il cui *iter* era già iniziato in Commissione ambiente del Senato, ha presentato al nostro esame un emendamento di contenuto analogo. Lo sottolineo: questa misura importantissima non è *ad personam*, ma la determinazione di questa anziana novantacinquenne ha consentito di portare alla luce centinaia di casi analoghi, di costruzioni temporanee costruite per far fronte all'emergenza del terremoto. Si tratta di costruzioni realizzate in autonomia da cittadini terremotati, soprattutto da allevatori e agricoltori che, non volendo o potendo lasciare la propria terra e il proprio luogo di lavoro, non potevano aspettare i mesi annunciati da Renzi, che poi si sono moltiplicati, per la consegna e l'affidamento delle SAE, le strutture abitative di emergenza. Un problema, quello delle casette, che per noi della Lega Nord è stato evidente fin da subito che sarebbe emerso. Lo abbiamo segnalato lo scorso anno

In un Paese dove l'abusivismo è diffuso e - ahimè - in gran parte tollerato, le Istituzioni devono applicare sempre il buon senso e comprendere le necessità di chi si trova, in una manciata di secondi, come in guerra, subendo devastazione, smarrimento, perdita di identità e, per anni, la permanenza in uno stato di assoluta precarietà, perché queste sono le conseguenze che portano i terremoti. La norma approvata, ormai nota come salva Peppina, è molto semplice. Non si tratta, cari colleghi del Movimento 5 Stelle, di una sanatoria tombale, prevede che per le casette costruite nelle zone terremotate l'attività sia di edilizia libera e ci sia la compatibilità paesaggistica, ma ovviamente a determinate condizioni: che il Comune appartenga al cratere del terremoto; che la casetta sia costruita in area di proprietà privata, con soldi propri in sostituzione di una SAE e, dunque, consentendo allo Stato di risparmiare non pochi soldi; che la casetta sia una struttura temporanea utilizzata a fini di abitazione principale. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Infine, che una volta terminati i lavori di ricostruzione dell'edificio danneggiato o distrutto, questa casetta venga rimossa.

necessariamente, a breve bisognerà tornare. Riteniamo sacrosanto che il diritto all'equo compenso debba essere riconosciuto a tutti i 2,3 milioni di professionisti con partita IVA e non solo a una categoria professionale. Infine, mi soffermo sulle misure nel campo della protezione cibernetica. bene che l'emendamento sia stato ritirato: la proposta di consentire alla Presidenza del Consiglio dei ministri la costituzione di una fondazione di diritto privato per la protezione cibernetica per attività di ricerca è, a nostro avviso, molto rischiosa. Noi pensiamo che la sicurezza cibernetica nazionale debba essere di dominio esclusivo di organi dello Stato e non allargata ai privati. Se proprio si ritiene che le agenzie AISI e AISE non possiedano le risorse e le capacità tecniche necessarie, che si faccia come in Gran Bretagna o negli USA, dove esistono agenzie dedicate. Permettere ai privati di entrare nel sistema di protezione dei dati è un rischio, perché possono esservi soggetti i cui interessi non necessariamente possono coincidere con quelli nazionali. Domando: che segnale dà al mondo un Paese il cui Stato appalta a fondazioni di diritto privato una parte sensibile della sua sicurezza?

di un provvedimento articolato che tocca tantissimi argomenti, sicuramente tutti importanti per il rilancio dell'economia del nostro Paese.

Siccome ci sono tanti interventi qualificanti, nell'azione emendativa ritengo che il Governo abbia dovuto subire anche delle angherie, soprattutto nel settore della sanità, ma non voglio polemizzare su questo aspetto.

uno dei tanti, a cui faceva cenno poc'anzi il collega Arrigoni, è quello delle Agenzie fiscali, rispetto alle quali il Governo ha presentato un emendamento che poi ha dovuto ritirare: forse, in certi casi, può anche essere meglio, perché fare un'ulteriore riflessione è importante, soprattutto perché noi del Gruppo ALA non condividevamo una serie di considerazioni di merito, in modo particolare

voglio poi dimenticare, perché per il nostro Gruppo è importante, che abbiamo fatto una proposta rispetto alla quale c'è stata una *défaillance* da parte del Governo e dell'intera Assemblea del Senato:

al relatore, il collega Silvio Lai, e in modo particolare al Governo, nella persona del vice ministro Morando, di aver compreso la concretezza dei nostri emendamenti e aver colto, con la sensibilità di sempre,

c'è stato qualche Ministro, qualche *leader* politico che ha promesso e si è impegnato, però nulla è stato fatto di concreto, neanche uno straccio di emendamento, mentre noi ci siamo ricordati, pur non andando a Ischia. Al di là di questo - non voglio avviare una polemica - condividiamo in linea di massima questo provvedimento, perché ha affrontato una serie di problemi

no. Per questo voglio ringraziare tutti i colleghi della Commissione, di maggioranza e di opposizione, che hanno contribuito

Signor Presidente, come scriveva pochi giorni fa un noto giornalista de «Il Sole 24 Ore», il decreto-legge di cui oggi discutiamo ha dato ampio spazio al manifestarsi di una «voglia matta di condoni e sanatorie» nella maggioranza, e aggiungerei anche di una voglia matta di condoni e sanatorie in quasi tutta l'opposizione; una voglia matta a cui assistiamo ormai da troppo tempo. tutte le fasi del prelievo fiscale, ad eccezione di quello che avviene alla fonte, prevalentemente sui redditi di lavoro e pensione, sono state oggetto di emendamenti con proposte di condoni e sanatorie: nessuna sanzione, nessun interesse di mora, e addirittura, in alcune proposte poi non approvate, nessun interesse *tout court* contro ogni ragionevole principio economico. Partiamo dall'avviso bonario: hai fatto una irregolarità, te la segnalo e puoi rimediare in sessanta giorni con una modica penalizzazione. Per chi non ha rimediato, è arrivata puntuale la proposta - poi non approvata - di sanatoria. Poi c'è la fase dell'accertamento: scopro che hai evaso e ti chiedo di pagare. Qui si aprono diverse possibilità: si è cercato, per fortuna senza riuscirci, di accorciare il tempo entro il quale gli accertamenti possano essere effettuati, con interpretazioni autentiche di norme esistenti, a favore di evasori già condannati e sicuramente noti a quest'Assemblea. A chi non ha pagato, è andato in causa, ha perso in due gradi di giudizio ed è giunto alla Cassazione, abbiamo dato, con provvedimenti recenti, la possibilità di salvarsi senza sanzioni, perché abbiamo rottamato le liti pendenti. In questo modo, alcuni grandi e noti contribuenti hanno risparmiato centinaia di milioni; centinaia di milioni persi per il gettito. Chi non ha pagato e non è andato in causa, ed è quindi arrivato alla fase della riscossione coattiva, ottiene una rateizzazione, che abbiamo riconosciuta, nella maggior parte dei casi, a prescindere dalla condizione economica: a prescindere, cioè, dalla difficoltà oggettiva che potrebbe avere a pagare le imposte. Per chi, poi, non ha pagato tutte le rate, ecco che arriva la rottamazione delle cartelle. Con il provvedimento, come emendato in Commissione con il sostegno di tutte le forze politiche, sono state eliminate tutte le barriere che ancora esistevano ad accedere a questa rottamazione. Non eri in regola con la rateizzazione? Vieni riammesso. Non hai versato nei termini tutte le rate della rottamazione a cui avevi aderito? Vieni riammesso. Questo è particolarmente grave, perché non c'è un condono (o sanatoria come la si vuole pilatescamente chiamare)

scomparire il patrimonio che sarebbe aggredibile con la riscossione coattiva. E intanto lo Stato perde gettito. L'innovazione più grave tra quelle introdotte con questo decreto-legge è che non si vanno a rottamare solo le cartelle vecchie, su cui ovviamente le pretese del fisco si erano affievolite, ma anche quelle nuove, di pochi giorni fa, per le quali le probabilità di riscossione sono invece molto alte. Perché questa rinuncia a priori? Stiamo dicendo che nonostante la tanto sbandierata riforma di Equitalia la riscossione non funziona? O che rinunciamo per principio a ogni attività di riscossione? Oppure stiamo dicendo che chi non paga le imposte deve sempre essere premiato? Riflettiamoci però: si tratta di un premio particolarmente ingiusto socialmente. Ricapitoliamo: un avviso bonario può segnalare un errore comprensibile che non significa necessariamente evasione. Chi, dopo l'avviso ha pagato nei sessanta giorni ha sopportato una sanzione, chi non ha pagato se la cava con nessuna sanzione e viene quindi premiato. Così per l'accertamento e la sua rateizzazione: chi sta pagando faticosamente ha la sanzione; chi non ha pagato non ha alcuna sanzione e lo stesso vale per la riscossione e la sua rateizzazione. Chi ha pagato faticosamente si è preso le sanzioni e chi non ha pagato se la cava con niente. Prendiamo anche la rottamazione: chi non ha pagato le rate previste doveva decadere dal beneficio e invece è riammesso. Anche in questo caso una beffa per chi si è sforzato e ha pagato. Quali sono le ragioni di questa orgia condonistica? Si dice per venire incontro alle imprese e ai contribuenti in difficoltà economica. Se così fosse sarei la prima a essere d'accordo, perché usciamo indubbiamente da una grave crisi economica, economica, e anche perché, in generale, nessun creditore ha interesse a strozzare il proprio debitore. Ma non è così: la norma è generalizzata e va a favore di tutti, indipendentemente dalla loro condizione economica. La realtà è che va a favore prevalentemente di chi non ha difficoltà economiche, di chi dispone di liquidità e cioè di chi può permettersi di pagare con la rottamazione rate più concentrate nel tempo e più alte rispetto a quelle della rateizzazione ordinaria. I contribuenti in difficoltà vengono usati come scudi umani per i grandi evasori, che guadagnano da queste misure non poche migliaia di euro, ma centinaia di milioni. Abbiamo casi celebri e il buco di gettito che ne consegue è enorme. Questa misura provoca un danno erariale che non è correttamente quantificato. Si preferisce incassare qualcosa subito invece che tutto il dovuto in un poco più di tempo. Inoltre tutti gli studi economici certificano che un condono oggi deprime il gettito di domani, abbassando il grado di fedeltà fiscale, perché ci si attende un nuovo condono e poi un altro e un altro ancora, com'è puntualmente avvenuto tante volte nel nostro Paese. Si dice che lo si fa perché le sanzioni sono eccessive, ma è stato questo Parlamento a riformarle solo nel 2015. Se non ci vanno bene cambiamole e non usiamole come scusa. Si dice che le sanatorie fanno emergere il nero e lo sradicano, ma nonostante siano state fatte ben due *voluntary disclosure*, nel solo 2017 la Guardia di finanza ha scoperto fatture false verso l'estero per 1,6 miliardi con 400 milioni di imponibile evaso. Anche in questo campo è stato messo a punto un nuovo condono: si tratta di un mini scudo che riguarda i transfrontalieri e gli ex residenti all'estero molto più generoso della *voluntary disclosure*. Infatti, chi ha fatto la *voluntary* perché aveva capitali di attività finanziarie all'estero non dichiarate ai fini del monitoraggio del monitoraggio aveva uno sconto sulle sanzioni, ma doveva versare tutte le imposte evase. Con questo condono invece si paga un piccolo *forfait* del 3 per cento del valore delle attività: un vero regalo. Le motivazioni portate per tutte queste sanatorie quindi non reggono. Io credo sia molto più importante quanto non si dice e cioè la verità. La verità è l'idea che le tasse siano comunque un furto e quindi meno le si paga meglio è. L'idea è che il contribuente deve difendersi da un fisco vorace che gli porta via ciò che è suo. Noi crediamo invece che il fisco sia lo Stato, che raccoglie risolse secondo regole decise democraticamente per finanziare i beni comuni per l'intera collettività e prima di tutto il *welfare* universale. Smantellare il fisco equivale a smantellare il *welfare* universale e a lasciare quindi che solo i più ricchi possano accedere alla sanità, all'istruzione, agli asili, all'assistenza ai più deboli, alla vita indipendente per le persone con disabilità. Le persone non pagano spontaneamente le imposte (si chiamano infatti imposte). Nel prelievo c'è un elemento coattivo che deve avvalersi, ahimè, anche di strumenti odiosi come i pignoramenti, a tutela però del benessere collettivo. L'evasione fiscale sottrae 100 miliardi e più all'anno al gettito, miliardi che in buona parte potrebbero essere utilizzati per ridurre le imposte a chi le paga fedelmente. L'evasione fiscale nasconde fondi per corrompere e finanziare illegalità, l'evasione fiscale intreccia con l'evasione contributiva, con lo sfruttamento di manodopera, con l'immigrazione irregolare e il caporalato. Va combattuta con determinazione, non continuando a riconoscerle dei premi. La rottamazione indistinta, la sua estensione ai ruoli appena emersi strizza l'occhio all'evasore e bastona chi ha pagato fedelmente. È un provvedimento indifendibile a cui noi ci opponiamo con forza.

Signor Presidente, signor Ministro, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi, prima di iniziare nel merito il mio intervento, devo riconoscere il lavoro svolto dalla Commissione e dal relatore, non solo per la complessità del provvedimento, ma soprattutto per le numerose revisioni ivi contenute. L'eterogeneità delle disposizioni che il Governo ha voluto affrontare in questa sede ha riguardato anche un tema a me caro: quello della produzione e trasformazione di *cannabis* a uso medico. Sono felice che il confronto sia stato libero da pregiudizi o posizioni di etica personale, un confronto pragmatico insomma, questo a dimostrazione della valenza - e della necessità - medica nella coltivazione della *cannabis*. Pur tuttavia, un appunto sul metodo mi sia concesso: avremmo potuto regolamentare meglio e con più coraggio la materia, soprattutto nel suoi aspetti più divisivi e delicati ma pur sempre rispettando e affrontando un tema che è ormai soprattutto di esigenza sociale. Regolamentare l'uso dei medicinali di origine vegetale a base di *cannabis* - nonché la sua distribuzione - è un dovere ancora più forte per noi legislatori perché dobbiamo dimostrare di occuparci del bene sociale con laicità e scevri da ogni pregiudizio. In particolare, le condizioni terapeutiche tratteranno casi di dolore cronico, soprattutto nei soggetti sottoposti a chemioterapia. Non possiamo permetterci, quindi, di rimanere indifferenti. Dico questo perché purtroppo il dibattito sulla liberalizzazione (nel testo approvato alla Camera e purtroppo non ancora calendarizzato in Senato) ha lasciato poco spazio all'approfondimento sull'uso medico,

oltre a quella già prodotta dallo Stabilimento chimico-farmaceutico militare di Firenze, definendo successivamente la natura giuridica delle strutture che eventualmente potranno essere autorizzate alla coltivazione e alla trasformazione, nonché eventuali controlli. L'importante è stato comunque stabilire la legittimità di questo passaggio, ovvero se il fabbisogno di farmaci e di materia prima evidenziasse gravi carenze nelle forniture rispetto alle richieste dei malati, si potrà avviare una produzione e un confezionamento in più siti. Sarà, poi, necessario un decreto del Ministro della salute per poter individuare i nuovi siti di produzione e rilasciare il nulla osta, siti di produzione che dovranno però operare rispettando le *good agricoltural and collecting practices* (GACP), ovvero secondo *standard* di produzione e di qualità definite dall'Agenzia europea delle medicine Non ritengo comunque ulteriormente rinviabile il tema della liberalizzazione della *cannabis* per uso personale. Anche in questo caso, con approccio laico e pragmatico, è necessario valutare come aprire a questa pratica anche nell'ottica della minimizzazione del danno, consci inoltre di poter così erodere i grandi illeciti guadagni che la criminalità organizzata ottiene. Questo però, temo, sarà valutato nella prossima legislatura. Durante l'esame del provvedimento, inoltre, in Commissione è stato purtroppo bocciato un mio emendamento che ho riproposto per l'esame dell'Assemblea sulla riduzione delle accise sulla benzina. Faccio una premessa, per chiarire meglio il termine della questione. Il Ministero dell'ambiente ha provveduto recentemente alla presentazione del Catalogo dei sussidi ambientalmente favorevoli e dei sussidi ambientalmente dannosi. Tale documento analizza tutti gli interventi fiscali in vigore che hanno un impatto ambientale classificandoli in tre categorie: i sussidi ambientalmente favorevoli, i sussidi ambientalmente incerti e i sussidi ambientalmente dannosi. Come sussidi intendiamo

sui carburanti da sole rappresentano un valore di circa 3,4 miliardi di euro. Una loro graduale riduzione e una riduzione delle esenzioni apporterebbe indubbi benefici sia alle finanze pubbliche sia all'ambiente. Per contro, il comma 1, punto 2, dell'articolo 5, nel modificare la lettera *c)* del comma 718 della legge di stabilità del 2015, stabilisce che l'aumento per l'anno 2019 delle accise sulla benzina e sul gasolio usato come carburante sia tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 10 milioni di euro, anziché di 350 milioni di euro. Il mio emendamento, pertanto, interviene sopprimendo il punto 2 del suddetto comma in modo da mantenere l'aumento già previsto.

tornano a crescere nel mondo le emissioni di CO2 (di anidride carbonica), come emerso durante la COP23 di Bonn, appena conclusa in questi giorni. Una cosa vorrei fosse chiara a tutti: per tutto ciò che approviamo in quest'Assemblea; per tutti gli interventi legislativi che mandiamo avanti, dovremmo valutare sempre attentamente il loro impatto sull'ambiente.

Presidente, questo che stiamo esaminando è un provvedimento che costituisce un segmento della manovra di bilancio. Non può sfuggire a nessuno che la manovra di bilancio che stiamo affrontando è quella di fine legislatura e non può sfuggire a nessuno che questo fatto implichi, sul piano politico, alcune considerazioni che si traducono poi anche in fatto normativo. Dico questo, signor Presidente, perché non possiamo estrapolare da un contesto sociale ed economico, penso anche politico e militare internazionale, questa manovra di bilancio, perché influenzerà bene o male, forse non in modo decisivo, anche il risultato elettorale. E le scelte che si fanno in queste ore non sono di poco conto, perché disegnano percorsi dare a questo Paese un destino positivo, un percorso di crescita e di sviluppo nella democrazia e nel rispetto delle istituzioni nate dalla Resistenza antifascista, oppure una deriva qualunquista autoritaria e restauratrice. Questo è il dato e non c'è nessuno che si possa lavorare le mani e liberare la coscienza da questo ragionamento, perché, se lo fa, è complice di quella deriva; se lo fa, aiuta quel processo di restaurazione. Anche questo provvedimento

di aver assunto un atteggiamento responsabile di fronte al Paese: non ci sono stati tentativi ostruzionistici, ostruzionistici, né conflitti pregiudiziali di tipo ideologico. C'è stato un tentativo vero da parte di ognuno di stare sul merito; un merito che non ha risolto tutto, ha lasciato grandi questioni di fronte a noi. a noi. Ci sono vicende che riguardano le persone, le famiglie, quelle che soffrono più di altre condizioni di difficoltà,

di disabilità, abbiamo ripresentato gli emendamenti in manovra di bilancio e penso che su tali questioni l'attenzione debba essere maggiore di quella che c'è stata fino ad oggi. Io ho sentito parole positive, l'annuncio di sensibilità che ritengo possano concretizzarsi prima della conclusione dell'esame della manovra di bilancio. Poi ci sono state questioni che hanno riguardato territori sofferenti, che sono state considerate; forse non tutte, ma molte sono state considerate in questo provvedimento. Penso a tutta la vicenda che riguarda i danni da terremoto, da calamità naturali, da emergenza climatica. Io stesso Io stesso ho avuto riconosciuto per la mia isola un contributo importante per il settore agropastorale, che da sempre è in sofferenza e che oggi ancora di più soffre una condizione di difficoltà proprio in ragione del cambiamento climatico, di periodi pesanti di siccità, di gelate inaspettate che riducono la capacità produttiva della terra e riducono pesantemente la possibilità di esistenza e di resistenza delle nostre aziende agropastorali.

stata un disastro, perché non abbiamo più la compagnia di bandiera e neppure una compagnia privata che si riferisca al nostro territorio nazionale, ma non è una responsabilità di questo Governo e neppure degli amministratori straordinari che sono stati nominati. Questa è una responsabilità antica, che ha radici nell'ingordigia dimostrata tanti e tanti anni fa e che noi non vogliamo ritorni. ragione facciamo una battaglia per l'unità delle forze progressiste e democratiche di questo Paese: non vogliamo che ritorni quel periodo.

rispetto ai pesanti ricordi, che ci trasciniamo, di situazioni certamente molto più negative e censurabili sul piano della produzione del diritto.

chiedo cosa avremmo dovuto dire negli anni in cui l'evasione fiscale a gogò veniva teorizzata da chi aveva le responsabilità prime delle istituzioni democratiche di questo Paese, il Governo e il Parlamento.

perché è un danno grave per il Paese, soprattutto per i lavoratori, le loro famiglie, coloro che vivono nelle periferie, quelli che non stanno bene, giorno affrontano la vita con la difficoltà della sopravvivenza, non con l'agiatezza di una vita gratificante. Noi riteniamo, che la manovra di bilancio, nel suo complesso, debba tenere in considerazione questo aspetto, anche sul piano politico. L'appello che rivolgo al Governo è di mettere tutta la sensibilità di cui è capace

Abbiamo di fronte una situazione pesante anche sul piano internazionale. Io provo a dire: facciamo uno sforzo; guardiamo le cose dall'alto. L'Europa è per noi qualcosa da salvare e anche un problema da gestire nella relazione con gli altri.

e ci impedisce di fare, tutto ciò che avremmo voluto fare, anche attraverso le norme che siamo in grado di approvare in questo Parlamento. Ci sono dei vincoli e, ogni volta che ci riuniamo con qualcuno che ce li ricorda, abbiamo un fastidio, però l'integrazione europea non si può interrompere per una violenta guerra di influenze per cui questo Continente si trova a Sud tutto il malessere, dal Medio Oriente al Nord Africa, che non fa altro che fare guerre e produrre fenomeni devastanti come l'emigrazione di massa dalla paura. Non può non tenere conto che tutto il confine lungo il Caucaso è in guerra,

Non si può non tenere conto che all'interno dell'Europa le identità disconosciute diventano un elemento deflagrante degli Stati nazionali e che gli Stati nazionali che si chiudono in se stessi finiscono per essere terreno di coltura delle teorie

tenere il Paese unito attorno a un progetto di sviluppo e crescita complessiva, che metta Nord e Sud insieme piuttosto che dividerli, quando dobbiamo fare questo, cioè ragionare, per esempio, sulla provvista finanziaria, ci sta anche che i percorsi messi in campo in modo articolato per contrastare l'evasione, per recuperare un pezzo di imposizione abbiano un senso, anche se non è il metodo che avremmo preferito.

falsate per assenza delle autorità competenti nel far rispettare le regole commerciali, il rapporto tra consumatore e impresa,

viziata dal pregiudizio o dalla strumentalità, non può diventare elemento di conflitto a prescindere. Ieri ho ascoltato un interessantissimo intervento su un punto, che cito perché riguarda il settore agricolo.

a presentare le certificazioni antimafia. Le certificazioni antimafia si fanno d'ufficio e vi provvedono le prefetture, che utilizzano le forze di polizia. Per verificare se uno è o non è mafioso, in ragione di 5.000 euro di contributo, noi avremmo ingessato tutte le prefetture e avremmo ingessato tutte le forze di polizia a cercare le certificazioni altrimenti non avremmo dato il contributo a quelle aziende agricole e a quelle famiglie di coltivatori. Da lì si è sviluppata una bellissima discussione sull'intoccabilità del codice antimafia. Se noi ci difendiamo dalle mafie in questo modo, signor Presidente, noi finiamo per consegnarci per pregiudizio politico proprio alle mafie. nuova finestra"). Salutiamo una delegazione del comitato Centro italiano femminile di Vasto, in provincia di Chieti, che sta assistendo ai nostri lavori dalle

fiscale, relativi a talune problematiche delle libere professioni e, più specificamente, degli avvocati. Tale categoria è stata oggetto di attenzione da parte del provvedimento in esame sostanzialmente in due punti. Il primo prevedeva, e ha raggiunto in gran parte il risultato, il risultato, l'abrogazione dell'obbligo assurdo e irragionevole di contrarre una polizza assicurativa antinfortunistica per la categoria degli avvocati, nonché

richiesto successivamente riguardo alle motivazioni della previsione di un obbligo antinfortunistico per una categoria che, pur con tutti i problemi che ha, non dovrebbe correre rischi particolari a livello fisico nell'espletamento della propria professione, ha rinnegato l'intenzione di voler obbligare gli avvocati a sottoscrivere una polizza antinfortunistica per sé. la circostanza che in Commissione bilancio è stato approvato - e di questo ovviamente dobbiamo ringraziare i colleghi di tutte le forze politiche - un emendamento del Movimento 5 Stelle che è riuscito ad abrogare quanto meno l'inciso contenuto nel secondo comma dell'articolo 12 della vigente legge professionale forense, all'obbligo di contrarre l'assicurazione. Rimane in piedi il resto di quella norma, che qualche problema di irragionevolezza, di coordinamento e anche di interpretazione temiamo continuerà a produrlo; sarebbe stato meglio abrogare l'intero comma in questione. risultato in termini di ragionevolezza. L'altro aspetto che ha interessato avvocati e liberi professionisti è stata la tanto attesa introduzione del principio dell'equo compenso, a fronte, come sappiamo, dell'ormai annosa abrogazione delle tariffe minime. In un periodo di crisi, come quello che stanno attraversando tutte le categorie professionali (quella degli avvocati è quella che conosco più direttamente) con effetti veramente sconfortanti, ci si aspettava francamente un intervento più incisivo e più chiaro nel voler introdurre un principio secondo il quale l'equo compenso delle prestazioni professionali dell'avvocato - e delle altre categorie professionali - fosse tutelato e mantenuto, a fronte del rischio, che sta diventando realtà, del precipitare di quanto disposto dalla nostra stessa Costituzione, che prevede una retribuzione per ogni tipo di attività lavorativa. Il risultato ottenuto dall'emendamento governativo è alquanto sconfortante e inefficiente, non coglie nel segno. Viene stabilito il principio

contrattuali contenute in queste convenzioni, che riguardano banche, assicurazioni e grandi imprese (poi vedremo come è stato esteso alla pubblica amministrazione), applicando un criterio di vessatorietà che comunque è facilmente aggirabile, con riferimento alle clausole elencate nel quinto comma, perché viene fatta salva la possibilità che dette clausole siano comunque operanti e non impugnabili qualora oggetto di specifica trattativa e approvazione. Personalmente ieri ho rappresentato in Commissione bilancio che si tratta di una norma facilmente aggirabile; infatti, a fronte di un contraente forte (la banca, l'assicurazione, la grande impresa), è facile trovare i modi per simulare una finta trattativa, una finta approvazione

Grazie

farle mandare giù alle centinaia di migliaia di avvocati e, probabilmente, di altri professionisti, che dovranno accettare, ad esempio, il fatto che le spese debbano essere anticipate a carico del professionista oppure la rinuncia al rimborso delle stesse. La sublimazione della follia è, poi, nella lettera *g)* del comma 5, in cui è previsto che «in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso di spese liquidate che siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte». Questo vuol dire, in sostanza, per chi non abbia chiaro il principio, che se la banca fa sottoscrivere una convenzione all'avvocato Castaldi

all'avvocato Castaldi rimangono 50 euro e la banca o l'assicurazione si arricchisce dei 450 euro di differenza. Siamo veramente alla follia. Ripeto: il tentativo di voler tutelare gli avvocati, a mio modestissimo modo di vedere, rischia di avere l'effetto esattamente contrario, perché sarà più difficile provare la vessatorietà delle clausole, essendo rimasto l'inciso «salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione».

qualora l'avvocato o il professionista volesse impugnare quella clausola avente un contenuto così vessatorio, ha un termine decadenziale di ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione. Capite bene che questo, nella gran parte dei casi, è un termine troppo ridotto e che parte quando la convenzione ancora deve esplicare i suoi effetti. L'estensione anche alle altre categorie professionali è avvenuta in maniera, noi riteniamo, raffazzonata, ma ci rendiamo conto onestamente, dal punto di vista intellettuale

che i risultati non saranno quelli attesi; dal nostro punto di vista c'è anzi il rischio che sia fatto ancora maggior danno alle categorie professionali, a quella degli avvocati in particolare. I medesimi emendamenti che abbiamo proposto, e che non sono stati approvati in questa tornata, saranno riproposti in sede di legge di bilancio e qualora, auspicabilmente, fossero ritenuti ammissibili, potranno essere l'occasione per la maggioranza e il Governo di un ripensamento e di un aggiustamento di questa normativa tanto attesa da centinaia di migliaia di partite IVA, che debbono fare i conti con l'ultimo taglio di *austerity* sancito dal Consiglio di Stato nell'ottobre del 2017, che ha stabilito che

per un bando proposto dal Comune di Catanzaro, con la sola soddisfazione dell'apparire esecutore di un progetto, pagato poi zero. Se mettiamo la pubblica amministrazione, anche a livello dei Comuni...

Auspichiamo che il Governo e la maggioranza vogliano concordare sui punti che abbiamo proposto negli emendamenti che saranno disponibili anche in tale occasione. Signor Presidente, onorevoli senatori, rappresentanti del Governo, sui giornali di oggi leggiamo due notizie che sembrano l'una contraddire l'altra. Da una parte, si riscontra il trionfalismo del Governo per le proiezioni ISTAT che danno un PIL in crescita all'1,8 per cento, la percentuale più alta da sei anni. Dall'altra, leggiamo la notizia che il vicepresidente della Commissione europea, rimprovera all'Italia per i conti non in ordine e anticipa l'idea di probabili provvedimenti da prendere nei confronti del nostro Paese, qualora non si registri una inversione di rotta già dalla prossima primavera. Sicuramente il PIL dell'Italia è cresciuto, non grazie all'azione del Governo, ma a causa di fattori esogeni. Mi riferisco, ad esempio, effetto Draghi, di cui più volte abbiamo fatto menzione nei nostri interventi in Aula, ed ora comprovato, in maniera empirica, dall'autorevole lavoro prodotto dal Centro studi «Economia Reale». Il prodotto interno lordo è migliorato e continuerà a crescere in funzione soprattutto della politica monetaria di Francoforte e del *quantitative easing* che vede la BCE acquistare titoli pubblici e che dovrebbe proseguire sino al terzo trimestre del prossimo anno, anche se con una intensità minore di quella adottata sinora. Così come sono ancora favorevoli le altre variabili esogene che hanno spinto la crescita della nostra economia, soprattutto il commercio internazionale e la stabilità del prezzo del petrolio. Anche le previsioni sulla crescita del nostro Paese sono conseguenti alle mutate variabili macroeconomiche. Ma ha certamente ragione il vice presidente Katainen: nelle manovre di bilancio italiane inviate a Bruxelles manca un serio impegno sui conti pubblici. La crescita italiana è largamente affidata al traino delle economie forti del mondo. Quasi nulla è stato fatto per ridurre la spesa, che anzi continua a lievitare, anche per effetto del decreto-legge in esame. Le coperture finanziare sono largamente affidate al *deficit* di bilancio. Lo *stock* del debito non solo non diminuisce, ma ha battuto i suoi *record* e temo ne segnerà di nuovi già dalla prossima primavera. In questo contesto si inserisce questo decreto-legge, che accompagna la manovra di finanza pubblica per il prossimo anno. Bisognerebbe dire per il prossimo triennio. In realtà, il lascito sugli anni successivi è solo quello di clausole poste a salvaguardia dei conti pubblici che prevedono aumenti delle imposte sui consumi, con un effetto depressivo sulla crescita. Da qui l'allarme, serio e documentato, della Commissione europea. Un provvedimento che, emanato per anticipare alcune poste sui conti del 2018, modificandole a partire dal 2017, rende però l'idea solo della provvisorietà degli interventi. Dopo l'esame della Commissione bilancio il provvedimento è quadruplicato nel numero di articoli, di contenuti e di interventi. Voglio sottolineare come dato di cronaca, ma molto indicativo,

che annuncia un disegno di legge di bilancio, di cui stiamo per iniziare l'esame, che potrebbe anch'esso lievitare nei contenuti visto il numero di emendamenti presentati dai colleghi. Troppi sono i problemi rimasti irrisolti durante gli ultimi anni, a cui si tenta di trovare una soluzione nello *sprint* finale della legislatura. Prendiamo, ad esempio, le norme sul sisma, che modificano i tempi e i modi della ricostruzione: interveniamo per la quarta volta in un anno su questo dramma. Parlo di dramma perché la gente del Centro Italia vive ancora in condizioni critiche e senza certezze sul futuro delle proprie case e attività.

Si introducono nel decreto-legge temi come la rottamazione delle cartelle, al solo fine di fare cassa e senza risolvere le tante questioni che riguardano imprenditori, professionisti e cittadini che non hanno potuto far fede ai propri impegni fiscali o contributivi, ma che intendono onorare i propri debiti con lo Stato. Insomma, si cerca di trovare una soluzione all'effetto tanto per fare cassa, senza pensare invece alle cause. Infine, per tornare agli effetti sui saldi di bilanci introdotti nella nostra premessa, voglio sottolineare che anche l'inserimento nel decreto-legge delle disposizioni che sterilizzano le clausole di salvaguardia hanno un effetto limitato. Fermando l'entrata in vigore delle clausole, non si riducono le tasse, ma si posticipano gli aumenti sulle imposte sui consumi, che scatteranno - purtroppo - dal 2019. Inoltre, come illustrato durante l'esame delle questioni pregiudiziali questa mattina, il decreto-legge contiene tutta una serie di disposizioni che sono presentate come urgenti, ma che in realtà cercano di affrontare situazioni irrisolte da troppi anni. Sto pensando, ad esempio, a casi come quelli della Croce Rossa, della bonifica ambientale del comprensorio di

Non era possibile pensare a un comparto mortificato nel compenso. Come abbiamo visto negli ultimi anni, i professionisti erano veramente alla mercé dei grandi gruppi e non riuscivano a fare quell'attività professionale che è importante per i nostri cittadini.

e di provvedimenti vessatori (mi sto riferendo allo *split payment* allargato) che, di fatto, contraddicono la volontà di andare incontro a garantire, con un equo compenso, un giusto riconoscimento dei professionisti che in Italia hanno fatto e stanno facendo tanto, anche in questi anni di grande crisi. Quindi, da un lato, un equo compenso e, dall'altro, un aumento della burocrazia. Siamo l'unico Paese che riesce a introdurre novità tecnologiche senza rimuovere alcun vincolo burocratico e questo credo sia davvero un grande macigno che lasciamo ai professionisti, ma - in generale - al Paese. Concludendo, si continua a mortificare il Paese, che non merita decreti-legge di questo tipo. Soprattutto, l'Italia non merita di avere un nuovo Esecutivo che si troverà, suo malgrado, di fronte a un futuro già ipotecato a causa delle scelte sbagliate adottate in questi anni dal Governo di sinistra.

penso che il dibattito che l'Assemblea ha sviluppato sia stato all'altezza delle aspettative che avevo in qualche modo evocato nel mio intervento. a tutti gli elementi che sono stati posti, perché penso che sia giusto concentrarsi su alcuni, in modo da poter dare delle risposte. Faccio una premessa. Penso che molto spesso noi diciamo le cose che servono, perché rappresentiamo delle parti questo ci impedisce anche di assumerci una responsabilità più ampia rispetto a quella che vogliamo soltanto rappresentare. questo per richiamare due delle questioni poste. Mi ha molto incuriosito e, in qualche modo, sono rimasto anche colpito dal fatto che sia stata presentata, da Gruppi che hanno avuto ruoli di Governo e che probabilmente avranno ruoli di Governo, una pregiudiziale di costituzionalità che, se fosse stata approvata, avrebbe generato un buco nel bilancio dello Stato equivalente

Non penso che qualcuno ci possa dire di essere una forza politica e una coalizione che pensa che questo sia un meccanismo stabile. In realtà, se non si prende atto del fatto che dieci anni di crisi economica possano aver generato una aver generato una frattura nel tessuto delle imprese, soprattutto delle piccole imprese e di quelle che si trovano nei territori più difficili e disagiati, e che questo abbia portato alla difficoltà

Questo non vuol dire che possa essere un meccanismo stabile, perché ha ragione chi dice che la fedeltà fiscale ha bisogno di certezze. Ma non possiamo - come d'altronde facciamo per i terremoti - non considerare che la crisi del 2008 è stata un terremoto sul piano sociale ed economico, con conseguenze evidenti. stesso modo voglio difendere e lasciare un segnale, affermando che ha ragione il senatore Micheloni, quando dice che risolviamo una questione del passato, con emigrati italiani, che sono già tornati in Italia e hanno somme all'estero regolarmente guadagnate e sulle quali hanno pagato tasse all'estero, ma oggi, se un lavoratore vive negli Stati Uniti per due anni, perché è un ricercatore universitario, si trova a pagare le tasse negli Stati Uniti e ad avere la difficoltà di riportare in Italia quello che ha guadagnato. Siccome siamo in un mondo che, sotto questo aspetto, è cambiato, perché il lavoro è cambiato, soprattutto per i profili elevati, è naturale che i cervelli vadano fuori ed è anche naturale che li riportiamo in Italia. Serve sicuramente affrontare questo tema in maniera definitiva e non occasionale e non soltanto - questo sì - con condoni all'indietro. Vorrei che il senatore Micheloni, quando vorrà tornare in Italia, non debba pagare ulteriori sanzioni e tasse in Italia, per cose che sono già tassate in un altro Paese, che tra l'altro ha regolari rapporti con il nostro. Penso Penso che dobbiamo prendere atto che c'è un cambiamento nelle abitudini dei lavoratori, che è più frequente di quello che pensiamo, tant'è vero che nel decreto-legge in esame, con una norma importante, abbiamo voluto restituire ciò che era anche in parte dovuto,

alla possibilità di estendere anche agli esercizi commerciali ciò che si fa oggi con la cedolare secca per gli affitti dei privati,

così come è politica per i piccoli Comuni, fatta qui - mi riferisco a chi ha detto che siamo stati distratti - la scelta di consentire, con una modifica della normativa, che le farmacie rurali

altri modi che rendono impossibile per le persone lavorare, non solo se c'è l'inagibilità, ma anche se ci sono danni gravi. Penso che la sua segnalazione dovrà essere consegnata alla 5a Commissione e al relatore al disegno di legge di bilancio, affinché il tema Ci sono danni che possono essere certificati, per esempio, dal commissario dell'alluvione, attraverso la Protezione civile, ed è giusto che l'alluvione di Livorno sia trattata trattata nelle modalità che consentono a quel Comune una ripartizione adeguata. Concludo ringraziando davvero tutti per il dibattito. Ci sarebbero state molte altre risposte da dare, ma penso che ci sarà un'ulteriore occasione per affrontare i temi segnalati.

Grazie